e che prevede interventi sia in materia tributaria che di sostegno alle imprese e alle famiglie, è composto da tre articoli. Nel primo, il Governo ha raggruppato una serie di proroghe cosiddette non onerose inerenti la stabilizzazione finanziaria, le proroghe riguardanti il trasporto pubblico locale (sia per i servizi di linea che per quelli non di linea)...

Si prevede inoltre un'estensione per il fondo di garanzia per la piccola e media impresa italiana, con la possibilità di accesso da parte delle imprese che si occupano di autotrasporto merci per conto terzi: un'iniziativa rilevante frutto della contrattazione avvenuta a livello nazionale con i rappresentanti del sistema dell'autotrasporto. È inoltre prorogato l'utilizzo dei *voucher* come sperimentazione per cassaintegrati e soggetti in mobilità. Inoltre, è stata prevista per alcuni settori che non sono coperti dalla cassa integrazione guadagni la proroga della cassa integrazione guadagni in deroga, una proroga per alcuni settori della magistratura, per i magistrati onorari e norme per l'emersione delle cosiddette case fantasma consistenti in fabbricati non accatastati o accatastati impropriamente al catasto rurale.

All'articolo 3, è prevista la copertura finanziaria di 93 milioni per il 2010 mediante il recupero da contabilità speciali, di 264 milioni per il 2011, una riduzione di autorizzazioni di spesa e reimpostazioni, e di 24 milioni per il 2012. Durante i lavori della Commissione, che sono stati intensi e costruttivi, grazie anche alla disponibilità

È stato reintrodotto ed esteso anche il meccanismo di esonero dal servizio per i dipendenti pubblici nei cinque anni che precedono il raggiungimento dei 40 anni di servizio, norma già presente presente nel nostro ordinamento per gli anni 2008, 2009 e 2010. Sono state previste, anche su iniziativa del Governo, una proroga degli sfratti

Ricordo inoltre che il Governo italiano è stato autorizzato a concedere garanzie per 766 milioni alla BERS, e questo permette alla Banca d'Italia, unitamente agli altri Istituti europei, di partecipare alle trattative per il prestito di 8,1 miliardi reso disponibile dal Fondo monetario internazionale.

BancoPosta, che svolgeva già una serie di funzioni di ordine bancario, ma con difficoltà nel settore dell'impiego non potendo svolgere tutte le funzioni. Con tale scorporo, il BancoPosta viene ad assumere le connotazioni di una vera e propria banca.

ricordare è ancora la possibilità per le società di assicurazione di valutare al costo storico e non al costo di mercato i titoli di Stato in loro possesso,

dell'editoria, delle televisioni, del FUS, degli enti locali, ed è stata prevista la possibilità di interventi anche di tassazione d'emergenza, con le addizionali o con un aumento dell'accisa sulle benzine, per le situazioni di emergenza territoriale a livello regionale. In ultimo, è stata permessa è stata permessa la sperimentazione della *social card* nei Comuni con oltre 250.000 abitanti per iniziative da parte di associazioni di volontariato. Sono rimasti inevasi tanti dei temi, tutti importanti, trattati dagli emendamenti dei colleghi, di opposizione e di maggioranza: i problemi affrontati dai 1.600 emendamenti che erano stati presentati in Commissione.

Il testo, tra le altre cose, fin dalla sua entrata in vigore, ha realmente reso possibile l'installazione del *WiFi* libero nel nostro Paese, consentendo perciò un'attività che che è molto importante per la comunicazione, specialmente per i giovani, ma non soltanto: ormai è diventato uno strumento prezioso di lavoro. Grazie al comma 19 dell'articolo 2, il *WiFi* è di nuovo libero

ne sono stati approvati ben 107, e questo è stato possibile grazie allo spirito di collaborazione che ha animato tutti coloro che hanno partecipato

sono stati approvati emendamenti che introducono il parere parlamentare sull'ulteriore proroga che il testo originale affida a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ripristinando un ruolo del Parlamento su questa fase; norme per un più razionale utilizzo dei rifiuti provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli; norme per agevolare il pensionamento di coloro ai quali manca poco per avere i requisiti per il collocamento con vantaggio per questi lavoratori e per la pubblica amministrazione; una norma per migliorare le garanzie di affidabilità sul rilascio dei brevetti di salvamento acquatico; una norma che razionalizza la proroga dell'impiego dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari; norme a favore della sicurezza nelle miniere; norme per un più razionale riscontro dell'idoneità alla guida dei ciclomotori (un fatto molto importante per la sicurezza stradale);

l'impegno alla futura corresponsione di queste parti restanti del trattamento di fine rapporto per poter concludere delle operazioni che probabilmente in molti casi si erano già impegnati a fare.

Ci sono delle norme per la ridefinizione del Programma della pesca e dell'acquacoltura, anche queste attività molto importanti nel nostro Paese. C'è una norma per favorire l'autosufficienza del nostro Paese nell'impiego degli emoderivati.

Voglio precisare che l'emendamento presentato dal relatore, approvato in Commissione, non toglie assolutamente nulla a coloro che si occupano di SLA, ma semplicemente evita che le somme che eventualmente questi enti non fossero in grado di usare, anziché

di quanto era destinato alla SLA, ma si fa sì che quanto eventualmente restasse venga usato per le finalità proprie del 5 per mille. È stata poi introdotta una serie di interventi a favore delle aree terremotate in Abruzzo, è stato prorogato per tre anni il meccanismo del *tax shelter*, che ha dato molto beneficio al cinema italiano, ma anche a

l'Italia è stata presente in diverse pellicole proiettate in tutto il mondo e prodotte non solo in Italia, ma anche in altri Paesi, è stato grazie a questo meccanismo, che viene prorogato fino al 2013. Vi sono poi numerose misure per la lotta all'evasione fiscale e misure e misure per la responsabilizzazione delle Regioni nella copertura dei costi della gestione del ciclo dei rifiuti. Vi è un intervento a favore delle autorità portuali; la razionalizzazione delle istituzioni scolastiche all'estero, un aspetto importante per la tutela della nostra cultura e della nostra lingua; vi sono norme per migliorare la cooperazione internazionale nel contrasto alla criminalità organizzata; la sperimentazione della carta acquisti a favore di enti caritativi. Vi è, inoltre, la sospensione della demolizione di immobili nella Regione Campania. Su questo, vi sono state polemiche e dichiarazioni. Si è parlato di incoraggiamento all'abusivismo edilizio, ma è semplicemente una norma che sospende per alcuni mesi la demolizione di immobili nella Regione Campania, ponendo un provvisorio rimedio alla situazione che si è determinata in quella Regione a causa di due ordinanze con le quali l'allora presidente della Regione Bassolino aveva

Corte costituzionale, ma nel frattempo tutti i termini erano scaduti, e di conseguenza si è creata la situazione alla quale l'emendamento approvato pone momentaneo rimedio. Vi sono poi interventi a favore dell'editoria e delle televisioni locali. Altro è stato approvato e non si può illustrare nello specifico, mentre è stato, come dicevo,

reso possibile: il presidente Vizzini, che ha guidato i lavori delle Commissioni, il presidente Azzollini, che sia come co-presidente, in quanto presidente della Commissione bilancio, sia come presidente della Commissione bilancio in sede consultiva, ha dato i pareri sugli emendamenti e su tutte le numerosissime riformulazioni, il collega relatore Pichetto Fratin, tutti i colleghi della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio, e anche i colleghi non appartenenti a queste due Commissioni che sono intervenuti per sostenere propri emendamenti o semplicemente per sostituire colleghi assenti. Infine, desidero ringraziare i consiglieri e il personale delle Commissioni che ci hanno coadiuvato in questo lungo lavoro.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, onorevoli relatori, ancora una volta (forse questa volta più delle altre) viene perpetuata la prassi di proroga di termini previsti dalla legislazione vigente il cui rinvio, o differimento, è reso necessario da ritardi o inadempienze delle amministrazioni pubbliche, in particolar modo delle amministrazioni ministeriali che dovevano garantire la fase attuativa delle leggi vigenti. questa è l'ennesima occasione in cui, a regolare cadenza annuale, o anche semestrale, si incide sul termine di entrata in vigore delle leggi per differirla o per prolungarla oltre il termine inizialmente stabilito, generando una crescente incertezza sulla qualità ed efficacia delle leggi mediante uno strumento normativo eccezionale che, per sua natura, dovrebbe essere temporaneo e tendenzialmente non ripetibile. La stessa eterogeneità delle norme contenute nel decreto‑legge in esame, appesantita

dicevo - ulteriormente appesantita dal fatto che sono state introdotte in Commissione 100 modifiche al testo

amministrazione, non rispettando i termini per gli adempimenti si propria spettanza, nell'immediatezza dello scadere ne dispone la proroga con proprio decreto, accrescendo così l'incertezza dei destinatari delle norme circa l'effettiva necessità di conformarsi ai termini scritti nelle leggi, in vista di continui e sistematici rinvii; C'è poi un aspetto particolare che sottolineo a lei, signor Presidente, e ai colleghi, che è totalmente innovativo. L'articolo 1 del provvedimento in esame è composto da due commi.

a ridosso del termine prorogato indubbiamente introduce una antagonistica concezione

tratta di un criterio totalmente innovativo, in quanto conferisce al Governo una sorta di delega che non è ammessa nella decretazione d'urgenza.

Oggi infatti siamo chiamati a valutare l'urgenza e la necessità di prorogare un termine, in linea con l'articolo 77 della Costituzione. come si collochi il rispetto di questo principio nel momento in cui deleghiamo il Governo ad introdurre un'altra proroga, ulteriore alla nostra, al

ossia stiamo innovando anche in materia del principio costituzionale che assegna alla decretazione d'urgenza determinati requisiti. Nel momento in cui si introduce una delega per prorogare ulteriormente, non potremo più valutare i criteri di necessità ed urgenza sui quali, invece, oggi siamo chiamati ad esprimerci. che tipo di controllo avremo nel momento in cui conferiamo una delega, peraltro discrezionale, al Governo per un'ulteriore proroga. Riteniamo che questo metodo innovativo rappresenti una violazione

il non passaggio all'esame del provvedimento, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, per violazione degli articoli 3, 76, 77 e 81 della nostra Carta costituzionale.

spostato e fatto diventare, con una tecnica che potremmo definire da OGM, regolamento a totale disposizione del Governo. Un gioco a incastro piuttosto pericoloso e illegittimo. Questo è il cuore della questione pregiudiziale.

Si può ritenere che un parere consultivo della Commissione parlamentare per la semplificazione o di quelle permanenti, comunque superabile dal Governo, rappresenti una seria riparlamentarizzazione e riesca ad evitare l'effetto Frankenstein? Evidentemente no. no. Aggiornando la pregiudiziale, segnalo altri tre problemi. Nel testo originario del decreto si riuscivano anche a prorogare quattro provvedimenti non scaduti

sembra anche che si voglia trovare lavoro da fare per le prossime legislature per il nuovo Ministro della semplificazione e per la nuova Commissione per la semplificazione. Infatti, scrivere una norma, come quella contenuta tutti «i termini e i regimi giuridici», eccetera, sono prorogati al 30 aprile 2012, eccetto gli altri, quando in realtà questa è una norma che vale solo per un caso, per le rappresentanze militari, è cosa piuttosto curiosa. Chi andrà a leggere la legge di conversione non capirà penserà di sbagliarsi, perché se si usa il plurale, parlando di tutti «i termini e i regimi giuridici», si penserà che i casi siano almeno due. Invece, questa norma «generale e astratta» è solo per la rappresentanza militare, ossia riguarda solo un caso. caso. Segnalo due altri problemi molto seri che, senza nulla togliere all'illegittimità complessiva di tale procedura,

non c'è una scadenza fissa o un termine preciso. Converrebbe pertanto scrivere che tali regolamenti sono da adottare entro il 31 marzo 2011, al fine di dare sicurezza ai cittadini sulla data di uscita dei regolamenti. C'è poi un ulteriore problema. La proroga ulteriore che si prevede è fino al 31 dicembre 2011, non al 31 dicembre 2011. 2011. Praticamente il Governo si troverebbe, caso per caso, con decine di proroghe, a stabilire termini diversi. Anche in questo caso, i cittadini si troverebbero in difficoltà nel capire quale regolamento viene emanato prima, quale dopo e da quando entra in vigore. Pertanto, sarebbe quanto mai opportuno stabilire che la proroga è al 31 dicembre 2011 e non fino al 31 dicembre 2011.

si vada contro quelle che sono state da sempre le segnalazioni e le direttive del Garante per la *privacy*, perché c'è il rischio che si ottenga una vera e propria

dei militari, abbiamo segnalato in più occasioni, anche con atti parlamentari che abbiamo depositato sia alla Camera, in particolare con l'onorevole Maurizio Turco, che al Senato, in particolar modo con il senatore Perduca, che tali proroghe sono davvero inaccettabili. Con il milleproroghe che stiamo esaminando è stata rimessa al Governo la possibilità di prorogare fino al 31 dicembre 2011 il termine di scadenza dei e dei regimi giuridici relativi a quasi tutti provvedimenti elencati nella Tabella 1. Tra questi, vi è quello relativo al mandato dei componenti in carica del Consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonché dei consigli centrali intermedi e di base dell'Esercito,

La circostanza che il decreto-legge in esame abbia un effetto non immediato assume rilevanza ai fini della valutazione circa la sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza.

(articolo 17, comma 3) prevede che: «Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie

delle garanzie previste per i regolamenti di delegificazione dalla legge n. 400 del 1988. Questa soluzione si pone nettamente in contrasto con il sistema delle fonti. Ho voluto intanto segnalare questi due ulteriori

In realtà, non ci sarebbe bisogno di argomenti a sostegno della nostra proposta di sospensiva: da una parte, si può fare la ricostruzione di questa incredibile vicenda della gestione commissariale del debito del Comune di Roma; dall'altra, esaminare il ruolo del Parlamento rispetto

ministri del 2008, che prevedeva una comunicazione trimestrale da parte dell'autorità commissariale dei flussi di cassa, degli incassi e dei pagamenti. Un'attività di monitoraggio prevista dall'inizio di tutta la procedura procedura di gestione straordinaria: anzi, una condizione e una garanzia, ovviamente, di controllo della stessa. L'atto di sindacato ispettivo e le lettere di richiesta formale non hanno però mai avuto alcun tipo di risposta. Andiamo avanti da un punto di vista cronologico ed arriviamo al

il 18 giugno 2010 dove quantifica il debito in circa 12,5 miliardi. Quindi, i miliardi salgono, crescono, si muovono, ma non si riesce ancora a capire effettivamente la cifra. A questo punto la conoscenza della documentazione aggiornata sulla ricognizione del debito e sull'attività di rientro dallo stesso appare assolutamente necessaria al Parlamento, proprio al fine di poter valutare le misure che sono contenute nel milleproroghe, in particolar modo al comma 7 dell'articolo 2, che concerne la proroga del termine dell'operazione di dismissione immobiliare, e all'ultimo capoverso del comma stesso, che incredibilmente cerca surrettiziamente di far approvare al Parlamento un documento di accertamento del debito che non è mai stato pubblicato e che lo stesso Parlamento non ha mai avuto modo di valutare. Noi, con la nostra questione sospensiva, chiediamo di sospendere il dibattito, di avere la documentazione e poi, in base ad essa, di poter fare le valutazioni e, quindi, di approvare

È la prima volta nei 150 anni dell'Unità d'Italia che il vertice amministrativo di un organo costituzionale dello Stato è ricoperto da una donna*.

La dottoressa Serafin ha ricevuto unanimemente stima e apprezzamento per la competenza, il merito assoluto, l'imparzialità, la dedizione al Senato e alle istituzioni repubblicane, dimostrati in tutti gli incarichi finora ricoperti. Verso tutti i Gruppi e i tutti i senatori il suo spirito di servizio è stato esemplare. Il suo impegno, la sua affidabilità professionale, la sua correttezza istituzionale sono nel solco di una grande tradizione e di una storia delle quali, senza distinzione di parte, possiamo essere orgogliosi. Storia e tradizione che abbiamo apprezzato nell'equilibrio testimoniato dal dottor Antonio Malaschini, presente in tribuna,

durante la sua lunga esperienza in Senato, prima di assumere il prestigioso incarico di consigliere di Stato, riconoscimento della sua fedeltà e del suo fondamentale contributo alle istituzioni del Paese. *(Vivi, generali applausi).* A lui e alla dottoressa Elisabetta Serafin i nostri migliori auguri di buon lavoro. Grazie*.

apprezzamento da parte del Gruppo di Futuro e Libertà. Credo che la nomina della dottoressa Serafin,

del Senato, quindi della seconda istituzione della Repubblica. Si tratta di un chiaro segnale di cambiamento culturale, una scelta che riconosce il ruolo delle donne in base alla meritocrazia e al rispetto

ha voluto calendarizzare in tempi celeri, ora all'esame in Commissione finanze e di cui sono relatrice, che prevede per la prima volta una norma di garanzia affinché nei consigli di amministrazione delle società quotate, nei collegi sindacali e anche nelle società municipalizzate almeno un terzo dei componenti sia sia del genere meno rappresentato, quindi, del genere femminile. È un importante provvedimento, anch'esso indice di un cambiamento forte. Alla dottoressa Serafin i nostri più vivi complimenti e auguri di buon lavoro. Volevo manifestare questo, perché non siamo presenti

la Presidenza coglie l'occasione del suo intervento, nel corso del quale ha ricordato di essere relatrice di questo importante disegno di legge che ci è arrivato dalla Camera dopo essere

sarebbe auspicio della Presidenza una calendarizzazione in Aula con un relatore, data la delicatezza del tema. Auspico quindi che attraverso il suo intervento da relatrice, e anche attraverso il senso di responsabilità di tutti i componenti della Commissione, questo testo possa arrivare al più presto in Aula.

grande professionalità, grande serenità, ma soprattutto grande imparzialità: una dote fondamentale per chi occupa un ruolo così importante. Sarà di ausilio a tutti noi, e a lei, Presidente. Quindi, complimenti, congratulazioni e buon lavoro, dottoressa.

che è stato emanato il 29 dicembre 2010 (parliamo quindi del lavoro svolto nelle Commissioni), rimarranno, signor Presidente, tracce abbastanza desolanti per la storia di questo Parlamento. Di che cosa sto parlando? LUSI). All'interno del decreto-legge, per le prima volta, si riconducono a norme primarie i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Si espropria il Parlamento della capacità di adottare norme primarie, sostituendole con atti del Presidente del Consiglio dei ministri. Su questo argomento e su altri, i nostri colleghi, nella Commissione affari costituzionali, prima, e poi durante il lavoro delle Commissioni riunite affari costituzionali e bilancio, sono intervenuti e hanno proposto soluzioni per risolvere il problema posto dall'articolo che nel decreto‑legge assumeva a rango di norma primaria i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Su questo argomento registriamo non solo che non c'è stata alcuna volontà di ascoltare le offerte di disponibilità alla soluzione di un problema, ma registriamo un pateracchio peggiore, signora Presidente, e cioè il fatto che alla una Commissione bicamerale per la semplificazione è stato assegnato il compito di esprimere dei pareri preventivi sugli schemi dei decreti legislativi che, a valle del decreto‑legge, delle norme del decreto-legge convertito in legge, dovranno essere emanati, previo parere delle Commissioni competenti per le questioni di carattere finanziario, cioè le Commissioni bilancio di Camera e Senato.

tappandosi le orecchie, la bocca e gli occhi. In realtà, il danno peggiore viene fatto dalla conclusione dell'emendamento approvato nelle Commissioni riunite che stabilisce che questi pareri sono di fatto ininfluenti rispetto al loro contenuto, perché laddove non intervenisse, oppure qualora non fosse conforme, comunque gli schemi dei decreti legislativi diventano norma vigente per il nostro ordinamento. Signora Presidente, questo è solo il primo dei passaggi di dubbia costituzionalità che hanno riguardato il disegno di legge di conversione del decreto-legge. Il secondo è ancora più drammatico per coloro i quali sono interessati, non certo al diritto, ma al modo nel quale questo Parlamento, in questa legislatura, forma il diritto e innova le legislazione vigente, ed è dettato da un emendamento presentato dai colleghi della Lega Nord nella giornata di martedì della settimana scorsa.

Che cosa c'è di strano o stupefacente in questo emendamento presentato venerdì? In fondo, si presentano emendamenti correttivi, o di sostegno, o di sistemazione che seguono l'argomentare del lavoro delle Commissioni riunite (in questo caso, affari costituzionali e bilancio). Magari, signora Presidente, sarebbe stato un lavoro costruttivo! Invece, questo emendamento presenta una strana modifica, non tanto alla legislazione vigente, signora Presidente, ma ad una sentenza della Corte costituzionale. Ebbene, venerdì della settimana scorsa, quattro giorni fa, una settimana dopo avere depositato - come tutti - correttamente gli emendamenti sottoposti all'attenzione delle Commissioni riunite, tre giorni dopo che i colleghi della Lega presentassero uno strano emendamento che riguarda i precari della pubblica istruzione in Italia, ci è stato presentato in Commissioni riunite un emendamento che, sostanzialmente, cita addirittura la sentenza della Corte costituzionale di poche ore prima per innovare, nel comma dell'emendamento, ciò che la sentenza della Corte costituzionale aveva stabilito in riferimento alla illegittimità di una norma che riguardava le liste dei precari della pubblica istruzione. Per coloro che ci stanno seguendo attraverso la televisione o attraverso la diretta radio stiamo discutendo di una piccolissima questione. Se si è iscritti nella lista di una provincia, per poter concorrere a fare delle supplenze in una scuola, o si è iscritti in quella lista, e allora si può sperare di essere chiamati,

nelle scuole di quella provincia, perché in quella lista non si compare. È un altro piccolo esempio di come i colleghi della Lega, sostenuti dalla maggioranza, pensano, ad esempio, il federalismo, di come immaginano la legittimità costituzionale di ogni lavoratore di questo Paese, che ha diritto di poter lavorare in ogni luogo di questo Paese. Se noi fossimo un Parlamento serio, questo emendamento lo avremmo visionato, discusso e poi ritirato mediante stracciatura. Invece no! Questo emendamento viene presentato, viene discusso, viene sostenuto dai colleghi della Lega nel silenzio dei colleghi della maggioranza, che, anche se non sono d'accordo con quello che c'è scritto, devono però sostenerlo per ovvi motivi di lealtà del Governo e della maggioranza a questa alleanza incredibile. Cosa andranno a dire i colleghi del Popolo della Libertà nelle Regioni del Centro-Sud quando qualcuno che li ha votati nel 2008 dirà loro di aver scoperto che hanno votato un emendamento che non gli dà la possibilità di andare a lavorare in una provincia diversa da quella della lista in cui è iscritto? Come verrà spiegata questa impossibilità? Non riesco ad immaginare, signora Presidente, che tipo di risposta potrà derivare dai colleghi del Popolo della Libertà. Sono però sicuro che nell'attenzione che essi prestano quotidianamente alle esigenze dell'elettorato saranno in grado di trovare una risposta chiara, precisa. Come non parlare, poi, signora Presidente, della grave violazione dei criteri delle leggi attraverso la palese violazione del procedimento di formazione di questo disegno di legge di conversione del decreto? decreto? Lei mi insegna, signora Presidente - come me lo insegna il rappresentante del Governo, autorevole esperto di diritto, oggi qui presente in rappresentanza del Consiglio dei ministri

quel parere era favorevole, signora Presidente, e all'unanimità le Commissioni riunite affari costituzionali e bilancio hanno votato a favore

è slittato il termine per far divenire condizione di procedibilità l'istituto della media conciliazione. Questo significa che ciò che doveva entrare in vigore il 22 marzo 2011 sarebbe entrato in vigore con molta più organizzazione, non solo logistica, da parte del Ministero della giustizia il 22 marzo 2012.

accaduto che, 24 ore dopo, un emendamento a firma del relatore ha modificato la norma di diritto sostanziale non modificata con l'emendamento del giorno Dal punto di vista formale l'emendamento era quasi ineccepibile, se non fosse che la violazione sta proprio nel fatto che l'ordine di presentazione per la votazione degli emendamenti da parte delle Commissioni riunite era stato falsato:

ma non avevamo mai visto una palese violazione nella formazione della legge all'interno di un procedimento legislativo nelle Commissioni di questo Senato. È stata, lo ripeto, una violazione palese. Signora Presidente, quando il giorno prima abbiamo votato l'emendamento all'unanimità, molti colleghi della maggioranza e dell'opposizione erano totalmente consapevoli di che cosa stessero votando, e non è, come dice qualcuno - e guarda caso, signora Presidente, non abbiamo sentito il Ministro della giustizia parlare di questo parlare di questo - che surrettiziamente i colleghi della maggioranza non sapessero che cosa stavano votando. Presidente, non approfondisco sul tema, perché se dovessi approfondire sul fatto che c'è un senatore - cosa alla quale non credo per principio - che è distratto e non si rende conto di che cosa sta votando, siamo un po' sul dramma, invece invece che parlare di cose serie. Quindi, parliamo di cose serie. Siccome molti della vostra maggioranza erano d'accordo con quella valutazione, cioè di rinviare di 12 mesi ulteriori, e ci sono pluri-testimoni in quest'Aula che possono confermarlo, anche oggi presenti e anche oggi assenti, voi in realtà, con l'ennesima sberla data di manrovescio sinistro, avete violato il rapporto tra Governo e Parlamento, inducendo le Commissioni riunite ad una sorta di sostituzione di se stesse rispetto al lavoro svolto la sera precedente, come se avessero dovuto rimangiarsi ciò che avevano legittimamente deciso. Per quale motivo? Il vero problema, Presidente, è che la sintesi del lavoro svolto dal Ministero della giustizia di via Arenula in questa legislatura è vicina allo zero: non c'è alcuna riforma portata a casa, non c'è alcuna modifica seria, a parte le cose che riguardano altri soggetti della pubblica amministrazione e che ogni tanto spostate dall'Interno alla Giustizia o agli Affari esteri, come se fossero sempre

Perché nell'organizzazione di questa nuova linea giurisdizionale, voi non siete stati in grado nemmeno di attrezzarla dal punto di vista logistico. Oggi il 65 per cento dei tribunali italiani non è in grado di dare uno spazio allo svolgimento della media conciliazione. Allora, cos'è stato fatto con quell'esempio? è stata approvata una norma che addirittura, per dare soddisfazione al ministro Alfano, ha anticipato l'entrata in vigore dell'istituto di circa 15-20 giorni, creando il famoso "spezzatino": alcune materie, perlopiù la maggioranza, entrano in vigore subito; altre, invece, diventeranno competenza di questo istituto nell'anno prossimo. nel maxiemendamento che il Governo porterà all'attenzione di quest'Aula - ancorché ciò non sia ancora ufficiale - per il voto di fiducia, cosa il Consiglio dei ministri abbia deciso di inserire su questo punto, così come su altri temi. Voglio andare verso la conclusione, signora Presidente, per parlare di tre temi, molto velocemente. Sulla base di un accordo unanime in Commissione, condivisa per il terremoto in Abruzzo. I più sanno che è una soluzione temporanea, cioè si è risolto il problema della mancata copertura da parte del Governo delle risorse necessarie per il posticipo della restituzione delle imposte sospese, provando a far sì che la norma che attualmente è stata approvata dalle Commissioni riunite risponda ad un termine infrannuale, e quindi non necessiti di copertura. È evidente che questo non è il provvedimento che risolve i problemi dei cittadini dell'Aquila e dei Comuni del cratere. del cratere. Noi del Partito Democratico auspichiamo (e lo abbiamo auspicato anche insieme agli altri colleghi delle Commissioni riunite non appartenenti al nostro Gruppo) che la prossima volta si trovi una soluzione definitiva. Abbiamo fatto proposte concrete, e sono all'attenzione del Governo: nessuno chiede cose impossibili. Sono tutte possibili dal punto di vista finanziario, e nel rispetto di un equilibrio complessivo. Se il Governo vorrà dare dimostrazione agli italiani che unanimemente si può trovare la soluzione al problema, troverà in questo Gruppo e nei suoi componenti un orecchio attento e una partecipazione seria. In ultimo, signora Presidente, segnalo l'incredibile distrazione - per essere eleganti sulla materia dei mutilati e invalidi del lavoro: un'attenzione distratta, perché fino all'ultimo momento c'era un'ampia disponibilità di tutti, cioè dei relatori e del Governo, a rispondere a problemi minimali. Signora Presidente, abbiamo visto che si è più capaci di risolvere il problema di come violare una sentenza della Corte costituzionale, piuttosto che quello di far fronte ai problemi dei mutilati e degli invalidi del lavoro di questo Paese.

si intrecciano in questo mille proroghe 2011 misure differenti ed il lavoro svolto è stato sicuramente positivo e dotato di una coerenza di indirizzo al punto che venerdì scorso il quotidiano «La Stampa» commentava: «Il provvedimento assume sempre più le sembianze di una nuova finanziaria». Io mi trovo leggermente in disaccordo

ma si orienta ormai il timone del Paese verso il mare aperto della crescita. In Commissione ho notato una certa condivisione trasversale su alcuni punti, malgrado le dichiarazioni di voto e le pubbliche prese di posizione; un atteggiamento che parla nei fatti, al di là delle dichiarazioni di facciata - come quelle che abbiamo appena sentito (il nostro collega sembrava un Orlando furioso del tipo «vorrei ma non posso», ma cosa doveva dire?) l'azione del Governo merita sostegno, specialmente, come accennavo, in un momento di svolta nell'approccio sui problemi della ripresa economica. Infatti, si sta attivando una forte azione di rilancio, dopo aver operato il contenimento del debito pubblico e della spesa dello Stato, con misure strutturali senza precedenti, perché era senza precedenti la situazione che si è dovuta affrontare. In questo contesto ritengo di particolare importanza l'approvazione dell'ordine del giorno che ho presentato in Commissioni riunite 1a e 5a insieme al collega Massimo Garavaglia, con il quale abbiamo chiesto al Governo di modificare e rendere flessibili i parametri di accesso al Fondo italiano di investimento per le piccole e medie imprese. Il livello di fatturato minimo richiesto (10 milioni di euro) esclude la gran parte delle piccole aziende in un momento economico estremamente difficile. È urgente per loro la rimodulazione del debito, magari causata dai ritardi nei pagamenti dei vari enti pubblici, insieme ad una forte patrimonializzazione; diventa vitale l'aggregazione e l'internazionalizzazione delle imprese per ampliare il *parterre* delle attività economiche di questo Paese. Portare a cinque milioni il fatturato minimo per l'accesso al Fondo consentirà di ampliare di qualche migliaio la platea delle aziende che potranno attingere agli oltre tre miliardi di euro di finanziamenti di cui è dotato il Fondo stesso, concorrendo al rilancio di vaste zone del Paese dove esse rappresentano le uniche attività economiche presenti, perché prima di farle aggregare e internazionalizzare, bisogna intervenire perché le stesse rimangano operative nel loro settore. Per converso, il tetto massimo consentito di 100 milioni di euro di fatturato, pur necessario come termine indicativo, a nostro avviso non andrebbe considerato rigidamente, perché diverse imprese superano di poco tale soglia e resterebbero così escluse dal conseguimento di obiettivi di crescita importanti per tutti, soprattutto in questo momento. Il Fondo italiano di investimento è uno strumento importantissimo per favorire lo sviluppo del capitale di rischio, lo stesso strumento utilizzato da tanto tempo da tante Nazioni del Nord Europa, che hanno seguito le direttive dell'Unione europea che prevedono proprio la aggregazione e la internazionalizzazione delle imprese. Esso, accanto alle nuove misure approvate nell'ultimo Consiglio dei ministri, può costituire il volano per rimettere in moto l'economia. La scelta del Governo di puntare in particolare sul sistema manifatturiero e produttivo, costituito dalle piccole e medie imprese, è una direttrice strategica che va condivisa e sostenuta con forza. È l'imprenditoria più sana e vivace che, se affiancata da uno Stato capace di *governance*, non certo di dirigismo, porterà nuova occupazione, nuova ricchezza e restituirà un ruolo internazionale e di prestigio all'Italia. manifestazioni di disapprovazione che abbiamo sentito su alcuni argomenti contenuti in questo mille proroghe, c'è stata una condivisione e ne abbiamo sentito un esempio prima dal collega. Mi riferisco alle norme per rispondere ai danni causati dalle alluvioni in Liguria, in Veneto, Campania e in Provincia di Messina; al rinvio delle imposte per i terremotati d'Abruzzo. Il recupero di queste imposte non deve essere troppo ritardato. Ve lo dico per esperienza: in Umbria abbiamo avuto dieci anni di ritardo nella restituzione della busta pesante. È stata una tragedia, prima e soprattutto per le imprese.

poi anche alla proroga degli sfratti per le categorie disagiate. Altre questioni aprono considerazioni più ampie di cui tener conto in futuro. Il tema del lavoro a tempo determinato nella pubblica amministrazione va affrontato in maniera nuova. Ritengo indispensabile un ribaltamento culturale: i Ministeri, le scuole e gli enti locali non sono ammortizzatori sociali. Se così sono stati considerati, allora è tempo che si cambi ottica. Ad esempio, a mio avviso deve far riflettere la conferma dei 650 lavoratori a tempo determinato delle questure, assunti nel 2002 per far funzionare gli sportelli unici dell'immigrazione al fine di affrontare quell'emergenza che, purtroppo, abbiamo visto proprio in questi giorni ripresentarsi ancora.

Nel decreto-legge in esame ci sono anche passi avanti che hanno faticato ad essere compresi e sui quali c'è stata un'esposizione mediatica negativa fortemente fomentata dall'opposizione. Mi riferisco al tema della fiscalità locale. Le Regioni si vedono assegnare la possibilità di incrementare le proprie entrate: possibilità, non obbligo. Su questo punto ci sono state tante prese di posizione incomprensibili,

L'opposizione si è scatenata anche con riguardo alla riapertura dei termini del condono edilizio del 2003 per la Regione Campania. La misura si riferisce ai soli immobili destinati a prima abitazione e permette ai cittadini campani di usufruire del condono statale

che aveva fatto prima il collega). Il provvedimento mira, inoltre, a risolvere l'annoso problema dell'emergenza abitativa nella Regione Campania, effettuando una revisione dei vincoli paesaggistici per giungere a una reale tutela del territorio. Credo sia giusto che i cittadini campani non paghino per le colpe della politica, perché quel condono venne recepito in tutte le Regioni. Concludo, sottolineando l'importanza politica dell'aumento dei fondi previsti con il cosiddetto 5 per mille, anche se resta la necessità di restituire maggiori risorse a un fondo che rende concreta l'autonomia dei cittadini nella distribuzione delle imposte. Siamo di fronte ad un atto di grande valore e che si ispira allo spirito liberale più genuino.

e l'incremento, seppur modesto, di 15 milioni di euro, per il Fondo unico dello spettacolo (poco conta quell'euro in più del costo del biglietto per andare al cinema). Credo, tuttavia, che in questo atto, che condivido e approvo, sia soprattutto sottesa una volontà politica forte che vuole ridare fiducia e prospettive di crescita al Paese, in modo da non adoperare più ammortizzatori sociali, ma creare posti di lavoro; non incentivi, ma opportunità vere per essere competitivi; non rigidità, ma meccanismi in grado di assicurare, nella flessibilità, il pieno utilizzo della forza lavoro. A questa volontà politica ritengo di non far mancare il sostegno di chi rappresenta la volontà popolare. PRESIDENTE. *(PD)*. Signora Presidente, nel processo di progressiva dequalificazione del bilancio pubblico e di costante peggioramento della trasparenza della gestione della finanza pubblica nel nostro Paese, questo decreto milleproroghe occupava un posto di assoluto rilievo già nella versione uscita dal Consiglio dei ministri. Cercherò di dare fondamento a questo giudizio attraverso due esempi, che saranno più che sufficienti. Innanzitutto, con il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge al nostro esame il Governo dispone, a furor di popolo, si potrebbe dire, data la gran messe di ordini del giorno parlamentari di destra, di centro e di sinistra che facevano voti in tal senso, il reintegro della somma necessaria a finanziare compiutamente il 5 per mille. Poiché il decreto-legge non contiene misure di aumento delle entrate, se ne deduce che la copertura finanziaria di questa disposizione debba essere ricercata attraverso risparmi. La copertura finanziaria di questa scelta invocata da tutti è ricavata in larga misura dalla riduzione delle somme disponibili per rimborsi e compensazioni,

stabilità - una volta chiamata legge finanziaria - il Governo sceglie di non finanziare le scelte dei contribuenti (quelle fatte attraverso la dichiarazione relativa al cosiddetto 5 per mille) a favore di associazioni, fondazioni e organizzazioni e organizzazioni *non profit*. Ci vogliono 350-400 milioni di euro e il Governo stanzia nella manovra finanziaria solo 100milioni di euro. Poi il Governo stesso, sensibile al sacrosanto grido di dolore che si leva a quel punto contro questa scelta assurda, prende circa 100 milioni di euro dei contribuenti (soldi che lo Stato è obbligato a restituire ai contribuenti perché hanno diritto a compensazioni fiscali e crediti di imposta)

Questa è la risposta del Governo Berlusconi scritta in questa legge (anche se nascosta alla comprensione dei più) che non arrivano mai. La risposta è la seguente: pazienza, hanno già aspettato tanto, aspetteranno ancora di più. Il bilancio, come è noto, è la sede che raccoglie le scelte allocative del decisore.

Eccola, dunque, la scelta allocativa del nostro Governo. Si prendono i soldi dei contribuenti che aspettano da anni che lo Stato paghi loro il dovuto e li si utilizzano per fare una cosa giusta, ma che non può essere finanziata in questo modo.

Il ragionamento del Governo e della maggioranza è stato di considerare che nessuno andrà nelle assemblee di artigiani, commercianti, imprenditori sull'orlo del fallimento perché lo Stato non restituisce loro ciò che è dovuto, mentre molti, da domani, andranno a pavoneggiarsi e a ricevere apprezzamenti per la soluzione del problema del 5 per mille. È sulla base di questo modo di ragionare sui problemi del Paese che si compie la scelta di cui sto parlando.

Un altro esempio da manuale di quello che non si deve fare se si vuole governare bene: il Governo, incapace di scegliere a chi dare e a chi togliere nel linguaggio dei bilancisti, di compiere la scelta allocativa di risorse scarse, costruisce con la legge di stabilità le condizioni per non scegliere affatto. Sceglie un bel fondo unico (750 milioni di euro) con dentro tutto e il contrario di tutto in termini di leggi da finanziare. Poi, lo stesso Governo, con il milleproroghe, usa quote rilevanti di quel fondo per nuove finalità che non sono quelle previste dalla legge di stabilità.

appena il Governo precisasse davvero di cosa si tratta, vale a dire rendesse chiara la scelta allocativa, la scelta di definanziare queste leggi risulterebbe politicamente insostenibile. Invece, al buio degli esiti puntuali della scelta, nessuno turba la quiete del decisore Governo. Vorrei contribuire a rendere questa quiete un po' meno tale, precisando di cosa si tratta. Con questa scelta, colleghi di maggioranza e colleghi del Governo, hanno molti meno soldi a disposizione,

il segno della crisi politica del centrodestra, la dimostrazione fisica della sua incapacità di scegliere tra istanze diverse, magari tutte legittime, attraverso l'esercizio dell'azione di governo fondata sul principio di responsabilità. Io mi prendo la responsabilità di decidere «a te sì, a te

fino a determinare scelte che fanno dubitare non solo della forza politica del Governo, ma dell'esistenza stessa di un soggetto che garantisca un qualsiasi indirizzo razionale

Da tanti anni, molti di noi sostengono l'urgenza di introdurre anche in Italia una qualche forma di assicurazione privata contro le calamità naturali. Assieme al professor Giarda, che considero uno straordinario Sottosegretario all'economia di quegli anni, elaborammo una proposta precisa, ispirata al principio solidaristico (ossia: i diversi territori, quelli più esposti al rischio catastrofale e quelli meno esposti, solidarizzino tra di loro) e e al principio di sussidiarietà (non faccia lo Stato ciò che può essere fatto dalla società: lo Stato intervenga quando e dove la società non è in grado e non è capace di intervenire). Demagogia e pressapochismo hanno impedito che negli anni si giungesse ad un qualche esito nella strategia di attuazione di tale riforma. Nel frattempo, abbiamo continuato a spendere sempre di più, sempre più male, sempre più in ritardo.

arriva una soluzione a cui nessuno aveva mai pensato, perché supera anche la fantasia: nessuno aveva mai pensato che si potesse fare una cosa simile. Secondo il Governo - udite, udite! - il modo migliore per uscire dal dramma di una calamità naturale consiste nel rifilare alle popolazioni colpite una vera e propria stangata fiscale: aumentare subito tutti i tributi, tutti i contributi e tutte le accise disponibili. Ciò è scritto nell'emendamento che presumibilmente verrà approvato domani da questa Aula nel maxiemendamento di fiducia. Verrebbe da dire: dopo il flagello di Dio le calamità naturali, per chi ci crede, le manda lui - segue il flagello di Cesare. Ho appena sentito la collega: federalismo anticatastrofe?

Vorrei essere chiaro. So che l'attuale situazione, aggravata dalla corruzione che ha sfregiato l'immagine pulita della nostra Protezione civile, è finanziariamente insostenibile: non possiamo andare avanti come abbiano fatto in questi anni. ciò bisogna porre rimedio con le riforme, non con le stangate fiscali. La ciliegina sulla torta, in questo contesto di irresponsabilità, la si trova nella norma sulle quote latte. Sull'aiuto diretto ai truffatori che ricattano la Lega e, per suo tramite, l'intero Governo italiano, è già stato detto tutto quello che bisognava dire. Anche a questo proposito, tuttavia, mancava la trasparenza della scelta allocativa, che è il tema di cui - come avrete capito - mi sto occupando. Ora, grazie all'emendamento approvato, tutti possono sapere quel che c'è da sapere: più 30 milioni - ecco la scelta allocativa - ai truffatori delle quote latte; meno 60 milioni, come da tabella fornita dalla Ragioneria generale dello Stato (per chi non ci crede, sappia che

Guardate, se tradirete l'impegno a rispettare il testo definito in Commissione perché togliete questo obbrobrio, noi vi capiremo e vi giustificheremo. La vogliamo dire così? Faremo uno strappo alla regola che vuole il rispetto alla lettera del testo uscito dalla Commissione da parte del Governo. Governo. In ultimo, vorrei fare un'osservazione di ordine ancora più generale. Signora Presidente, i nodi, quelli del Paese, stanno giungendo al pettine. In Europa si sta scrivendo il nuovo Patto di stabilità e di crescita. Il Consiglio europeo di marzo sarà decisivo. I nuovi *stress test* delle banche sono imminenti. Se ne è già decisa la qualità, e sapete che sono molto diversi da quelli che abbiamo brillantemente superato nel recente passato, tant'è vero che quelli non individuarono la situazione di esposizione, che le ha portate al fallimento, delle banche irlandesi. i prossimi sono una cosa seria. La crisi del debito sovrano in Europa non è superata.

Su tutto questo, nei prossimi giorni, dovranno essere prese decisioni destinate a influenzare durevolmente il nostro futuro, ben al di là di questa legislatura. Il Governo vuole decidersi o no a rivolgersi al Paese con un linguaggio di verità per sollecitarne l'impegno consapevole alla soluzione

Noi diciamo: «dimettetevi e andiamo a votare». Meglio il voto che una situazione di questo tipo! allora fatevi carico dei problemi del Paese. In questo provvedimento non l'avete fatto, anzi li avete aggravati tutti.

il titolo del disegno di legge oggetto di questa nostra discussione generale «Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie».

Ma al di là della battuta, di cui chiedo perdono, parto dalla seconda parte del titolo e dall'accenno, che io ritengo importante, cui faceva riferimento il collega Morando due minuti fa. La seconda parte del titolo dice: «interventi urgenti in maniera tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie». Già questa parte del titolo potrebbe essere condivisa, partendo da un'analisi: siamo di fronte ad una situazione economica e sociale oltremodo seria e difficile, contrariamente a quello che è stato detto in

e che adesso ci saremmo avviati ad una ripresa. Purtroppo così non è. La situazione, fuori da questa Aula, nelle case delle famiglie, nelle decine di migliaia di piccole e medie imprese che stanno morendo come mosche, è molto seria. E quindi credo di dover richiamare l'attenzione di questa Aula e del Governo ed anche delle opposizioni sul dovere civico che dovremmo sentire tutti, oltre che sulla responsabilità politica di affrontare questo tema. Ovviamente non ci si può più dire che il milleproroghe non può contenere manovre di politica economica, visto che lo scorso anno nel milleproroghe è stata fatta una manovra di politica economica per decidere come spendere i miliardi incassati con lo scudo fiscale per il rientro dei capitali: quindi, non esiste più l'argomento di incompatibilità della materia; allora il tema non è più formale, cioè valutare se in questo provvedimento è possibile costruire una vera manovra di politica economica. urgente - credo che la situazione lo dimostri di per sé - una manovra di politica economica. È urgente per affrontare la situazione delle famiglie e delle imprese, per sostenere la crescita, lo sviluppo, ma è urgente anche perché, come ricordava il collega Morando, a marzo il Consiglio europeo darà le nuove linee. Là non possiamo certo scherzare più di tanto. I colleghi ricordano - spero - tutte le mie annotazioni critiche verso questo eccessivo potere burocratico delle istituzioni europee. Ma io ho sempre distinto questo mio giudizio politico sull'assetto europeo dalla necessità addirittura di pensare il più rapidamente possibile agli Stati Uniti d'Europa, cioè all'entità politica europea, unica sede dove può esserci un futuro per l'Italia e per l'Europa nel nuovo mondo della globalizzazione.

a sostegno delle famiglie; delle imprese, della ricerca, delle infrastrutture e delle forze di sicurezza: altro che tagli orizzontali che magari vanno ad incidere sulla benzina dei carabinieri! Come di consueto, abbiamo indicato con nome e cognome le voci di spesa, corrente e non, che, nei nostri emendamenti, proponiamo di tagliare in modo molto forte, anche se modesto rispetto all'entità complessiva di quelle voci di spesa, per ottenere le risorse che potrebbero essere immediatamente messe a disposizione come sostegno alle famiglie, con le deduzioni per carichi di famiglia, quello che volgarmente viene chiamato coefficiente familiare; alle imprese, con il taglio

con 3-4 miliardi veri per la modernizzazione infrastrutturale del Paese, con 2 miliardi per la ricerca e l'innovazione tecnologica e con un miliardo per le forze di sicurezza. Quella manovra di politica economica che avevamo presentato nel corso della finanziaria per il 2010; finanziaria per il 2010; quella stessa manovra che il Governo ci chiese di trasformare in un ordine del giorno; quella stessa manovra che che il Governo fece propria accettando l'ordine del giorno. Quindi, la domanda è molto semplice e banale: essendo passati 14 mesi dall'impegno preso in quest'Aula dal Governo di seguire quelle linee di politica economica, noi vogliamo fornire un'ulteriore occasione. In questo milleproroghe quella manovra c'è: ci dica il Governo se intende o non intende farla; se non intende farla, viene meno all'impegno assunto in quest'Aula quando fece proprio quell'ordine del giorno. Ma proprio per agevolare la valutazione, l'analisi, la meditazione, sulla decisione da prendere (che come ormai sappiamo sarà presa attraverso il maxiemendamento sul quale il Governo porrà la fiducia, e quindi l'auspicio è che dentro quel maxiemendamento ci sia una decisione coerente da parte del Governo di rispettare l'impegno preso in quest'Aula nel dicembre 2009 e di cominciare a percorrere quella strada di politica economica vera) come ho già avuto modo di dire, sono aggiuntive rispetto alla necessità di mantenere sotto controllo i saldi finanziari. Queste proposte migliorano i saldi finanziari, sostengono la crescita, l'occupazione, la competitività, la ricerca, l'innovazione, l'università; e sono atti concreti, certamente molto più concreti e molto più rapidi da assumere che non una fantomatica revisione dell'articolo 41 della Costituzione che, ammesso che possa essere una componente di un'eventuale politica di sviluppo e di scossa all'economia, ha un tutti - che si completerebbe alla fine del 2012; ed eventuali effetti di una modifica costituzionale che preveda che è lecito tutto ciò che non è proibito personalmente li potrei quantificare in uno 0,1-0,2 per cento E allora, domani, dopodomani, c'è una cartina al tornasole. Se veramente il Governo, come credo debba fare, di fronte alla situazione economica e sociale che abbiamo, al di là degli slogan e della propaganda, fa proprio ciò che ha assunto come impegno in quest'Aula e decide, domani, di fare politica economica, farà cosa ben diversa dal dovere di salvaguardare i saldi finanziari. Quello è un dovere d'ufficio, un atto dovuto: non è la politica economica! Non vorrei usare il termine tecnico, ma molto appropriato, che ha usato il collega Morando: la politica economica è quella che decide l'allocazione delle risorse, non quella che fa *deficit* e debito pubblico. La politica economica è quella cosa in cui la politica si assume la responsabilità di dire: da quella voce, da quel capitolo, tolgo dieci perché vado a metterlo, magari solo per otto, in quell'altro capitolo, ed eventualmente il due di differenza lo utilizzo per ridurre ulteriormente il *deficit* pubblico.

con un filo di speranza, che non deve mai essere perduto) presentato come contributo a questo provvedimento, anche collegandoci alla seconda parte del titolo che reca Per agevolare l'analisi del Governo, queste nostre proposte le abbiamo divise in tre diversi emendamenti. Il primo emendamento è quello complessivo. Una manovra - non si spaventino i colleghi - di 35 miliardi di euro, appena appena il 2 per cento del prodotto interno lordo: è ora di finirla di presentare manovre dello 0,01 per cento del PIL e dire che sono manovre di sostegno all'economia. una manovra di dimensioni quantitative relativamente consistenti: 2 per cento del PIL è molto meno - quasi la metà - della manovra fatta dal Governo Amato nel 1992, almeno inizialmente stimata in 90.000 miliardi di vecchie lire, ma enormemente meno difficili di quelle che dobbiamo affrontare in questi giorni e in queste settimane. Da qui il richiamo alla responsabilità politica del Governo, della maggioranza e anche delle opposizioni. Noi interpretiamo la nostra responsabilità nel modo che sto dicendo, cioè proponendo azioni di politica economica che, peraltro, se fossero state fatte un anno e mezzo fa forse avrebbero oggi determinato una situazione economica e sociale nel Paese, non certo rose e fiori, ma un po' meno difficile di quella che appare, a parità di saldi finanziari, con il rispetto più fermo di quello che in gergo si chiama il rigore finanziario. per agevolare l'analisi, abbiamo diviso questa nostra proposta in tre stadi. Il primo stadio è quello che auspichiamo (visto che si deve fare, tanto vale farlo sul serio),

della politica economica italiana e della finanza pubblica: il bubbone che inquina il rapporto tra economia e politica, tra finanza e affari e cosche mafiose. Quelle due voci alimentano i flussi criminali. Il grande merito del ministro Maroni è stato quello di aver avuto importantissimi risultati anche in termini di sequestro dei patrimoni dei mafiosi. Ma se stimiamo il sequestro dei patrimoni in 20 miliardi di euro, dobbiamo sapere che quello è uno *stock* di patrimonio, mentre con il bilancio delle pubbliche amministrazioni noi alimentiamo, con un flusso annuale di 30‑40‑50 miliardi all'anno, quegli stessi patrimoni. Quindi, sequestriamo meno della metà in termini di *stock* di ciò che diamo come flusso ogni anno. Questo è lo scontro-confronto politico, perché una volta affrontato il taglio di queste voci allora è più facile poter concordare sulla distinzione di quelle risorse: alle famiglie, alle imprese, alla ricerca, alle infrastrutture. Proprio per questa ragione abbiamo voluto dividere in tre parti. Innanzitutto, un emendamento complessivo; poi, un emendamento di dimensioni più ridotte e forse più prudenti. Vogliamo cominciare a tagliare quelle due voci di spesa-bubbone in modo più prudente? l'entità complessiva è di 35 miliardi, cominciamo a farne almeno la metà facendo partire le agevolazioni alle famiglie, alle imprese e a tutto il resto con dimensioni più contenute.

il monte salari. Si potrebbe partire almeno con queste due piccole gambe, per poi procedere magari, negli anni successivi, con ulteriori tagli di spesa e con l'ulteriore rafforzamento del sostegno alle famiglie e alle imprese, estendendo le deduzioni per carichi familiari ad importi via via più elevati e il taglio dell'IRAP ad imprese con un numero di addetti via via più elevati, oltre il primo modulino dei 50 addetti. Ecco, signora Presidente, questo è il nostro contributo positivo. Il Governo nei giorni scorsi ha detto che c'è bisogno di un rilancio dello sviluppo; il dibattito in corso finalmente pare - almeno negli *slogan* essersi indirizzato anche al sostegno della crescita, delle famiglie e delle imprese, tanto che è scritto nel titolo di questo provvedimento. Certamente, però, non sono gli *slogan*, il fumo negli occhi dell'articolo 41 della Costituzione, che possano incarnare un senso doveroso di risposta al Paese in termini di politica economica vera. Un ultimo accenno infine, signora Presidente. A marzo si terrà il Consiglio europeo. Abbiamo di fronte Basilea 3. Non so se tutti sono consapevoli

diventano devastanti per il sistema economico e produttivo italiano. Nello specifico, applicare in modo automatico i nuovi parametri di patrimonializzazione delle banche significa che nei prossimi mesi vivremo un'ulteriore strozzatura del credito, mentre stiamo parlando di sostegno della ripresa. della ripresa. Si ventila che nel maxiemendamento il Governo intenda - a mio parere positivamente - inserire la possibilità inserire la possibilità per il sistema bancario italiano di utilizzare parametri europei anche in termini di valutazione dei pezzi di patrimonio che ancora oggi non possono emergere per far emergere il vero patrimonio del nostro sistema bancario in modo da poter rispondere alle nuove regole europee con più patrimonializzazione, facendo emergere una valutazione più corretta delle partecipazioni, delle sofferenze e quant'altro. Questa, eventualmente, è la parte positiva di un provvedimento ventilato in quel senso.

una riforma profonda, strategica del sistema Poste e di BancoPosta? Se c'è bisogno, come c'è bisogno, di una riforma strategica, strutturale di BancoPosta, credo non sia il decreto-legge

Non si tratta semplicemente di un fatto tecnico, ma di un fatto profondamente politico: stiamo parlando, infatti, del destino del risparmio di milioni e milioni di poveri cristi italiani che, come sappiamo, affidano al sistema postale la difesa del loro risparmio. Sull'utilizzo di quel risparmio, che è appetibile da mille parti, in Italia ed in Europa, il Parlamento dovrà esprimere una sua valutazione, doverosa da parte del Governo, in termini di piani strategici, di motivazioni strategiche, di piani industriali, perché una riforma importante come quella di BancoPosta possa essere attentamente valutata. È una

*(LNP)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, l'argomento all'ordine del giorno, che vede impegnate da qualche settimana tutte le forze politiche, non si deve prestare a facili strumentalizzazioni o ad interessi di parte. È stato, sicuramente per noi della Lega Nord, un momento di verifica, messa a punto, approfondimento di diverse questioni aperte e bisognose di definizione o di maggiori tempi per risolverle. La Lega Nord, naturalmente, ha a cuore le esigenze dei territori del Nord ma, come ha sicuramente dimostrato nei lunghi lavori di Commissione, anche l'interesse generale di tutto il Paese. Un argomento che mi è stato particolarmente a cuore - e voglio citarlo in questo mio breve intervento - è quello che riguarda tutti i lavoratori che si trovano a dover affrontare il problema delle controversie in materia di lavoro dinanzi la Corte di cassazione. Con il recepimento del nostro emendamento anche per quest'anno si evita l'applicazione del nuovo contributo unificato, che ovviamente avrebbe pesato sulle tasche del lavoratore. Va evidenziato, infatti, che l'introduzione di tale contributo rischierebbe di disincentivare la piena tutela giudiziale del lavoratore. Altro argomento a me caro, in quanto "laghée", riguarda la navigazione interna dei nostri laghi. Per ora abbiamo evitato il danno; dobbiamo trovare una soluzione definitiva in quanto è dal 1997 che si parla di regionalizzazione della navigazione dei laghi, che è la soluzione che può rappresentare la svolta purché naturalmente alle Regioni arrivino le risorse necessarie per portarla avanti. Noi sappiamo che la Regione vuole avere la certezza di prendersi in carico un servizio insieme ai fondi necessari per farlo funzionare meglio. Con il nostro emendamento siamo intervenuti anche sulla navigazione dei laghi, come il Garda, Como e Maggiore, consentendo l'utilizzo di risorse proprie senza incidere sulla finanza statale se non, con un nostro specifico emendamento, per due milioni, nell'ottica però che nel prossimo futuro le Regioni non debbano sempre andare con il cappello in mano fino a Roma e possano decidere loro come affrontare la questione senza dipendere da risorse Ricordo ancora come nel 1999 l'operazione di trasferimento alle Regioni, avviata dal Ministero dei trasporti e della navigazione, non fu perfezionata in quanto lo Stato non mise a disposizione delle Regioni interessate - Lombardia, Piemonte, Veneto - e della Provincia autonoma di Trento le risorse necessarie al rinnovo della flotta e al funzionamento del trasporto su lago, come espressamente previsto per legge. ricordo infine che nel 2006 la Regione Lombardia ha riattivato un nuovo confronto con le istituzioni regionali, costituendo un tavolo tecnico con la collaborazione di Ferrovie Nord Milano. Questo ed altro hanno sicuramente migliorato il testo iniziale, nella speranza che questo provvedimento, alla fine, consenta a questa macchina Paese di proseguire un cammino con qualche ostacolo in meno. A proposito di quote latte, mi consenta un'ultima battuta, signora Presidente. Io non so chi sono i truffatori o chi sono i truffati, ma, caro senatore Morando (che non è più presente in Aula), questo lo lasci decidere a chi dovrà giudicare, visto che ci sono delle indagini in corso.

il decreto di proroga termini quest'anno si caratterizza per una particolare eterogeneità e complessità delle materie e si caratterizza anche - credo molto negativamente - per un'assoluta illeggibilità delle norme in esse contenute; tutto questo alla faccia della semplificazione e della trasparenza più volte declamate. Soltanto per comprendere la materia di cui si sta trattando, si deve fare una specie di corsa ad ostacoli, avendo a disposizione il complesso della legislazione vigente, per individuare passando da norma a norma di quale materia si tratta. Considerato questo carattere, che a mio avviso è molto negativo, reputo non condivisibile dal punto di vista politico, oltre che dal punto di vista giuridico e della costituzionalità, la norma

c'è un'ampiezza di contenuti di rilevanza politica molto grande, ma dall'altro c'è un sovvertimento della scala gerarchica delle fonti del diritto, laddove si espropria il Parlamento dalla possibilità, che è giuridicamente rilevante, di intervenire sulla proroga di termini legislativi: si modificano leggi attraverso decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Ritengo questa scelta di assoluta gravità. Entro nel merito di alcuni temi, in particolare riferendomi alle materie della scuola e dell'università.

che è assolutamente contraddittoria ed irragionevole e pertanto incostituzionale. Mentre si discuteva del tema, che la maggioranza ha voluto introdurre in Commissione, del reclutamento del personale docente e delle graduatorie di riferimento che riguardano centinaia di migliaia di persone, è stata pubblicata la sentenza n. 41 del 7 febbraio 2011 della Corte costituzionale,

La norma che la Commissione ha approvato dice sostanzialmente questo: vengono bloccate le graduatorie degli insegnanti fino al 30 settembre 2012, quindi per il prossimo anno scolastico, facendo però naturalmente salvi gli effetti

di migliaia di persone, che sarebbero state messe in ruolo in modo improprio e quindi la sostituzione di queste persone con altre che invece erano collocate in fondo alla graduatoria, non è possibile non rifare le graduatorie.

ogni anno da persone magari differenti, ma che hanno un incarico annuale e che quindi hanno lo stesso costo di una persona immessa in ruolo e stabilizzata. La soluzione è utilizzando tutto questo consistente gruppo di posti liberi nel prossimo anno scolastico, in modo da risolvere positivamente il caos che si è determinato per la protervia del ministro Gelmini, che ha insistito nel voler dare applicazione a norme che già vari tribunali amministrativi avevano giudicato illegittime; una protervia che ha portato ad approvare l'articolo 1, comma 4-*ter*, come una sorta di sanatoria, perché già i tribunali amministrativi avevano proposto il commissariamento. Chiedo quindi da un lato il blocco della norma approvata in Commissione e dall'altro un piano di

il merito degli studenti che hanno ottenuto 100 o 100 e lode agli esami di maturità e una media alta nell'ultimo triennio di scuola.

Signor Presidente, il decreto-legge n. 225 del 2010 si presenta come un provvedimento particolarmente disorganico. Certo,

questioni pregiudiziali, si fa qualcosa di più: si adotta una tecnica legislativa che differisce da quella che ha caratterizzato i precedenti decreti milleproroghe. Infatti, tali decreti, senza modificare formalmente la disposizione vigente, disponevano la proroga della sua efficacia temporale.

una novità davvero rilevante, che permette al Governo una discrezionalità di proroga prima non consentita, che va al di là delle ragioni di necessità e urgenza. Come se ciò non bastasse, si preannuncia l'ennesimo voto di fiducia: un voto di fiducia su un testo maxiemendato e dai contenuti largamente insoddisfacenti. Non basta certo aver accolto nelle Commissioni di merito alcuni emendamenti dell'opposizione per cambiare il disegno di questo provvedimento, anche se è sicuramente da apprezzare l'accoglimento dell'emendamento che prevede che l'applicazione delle disposizioni del collegato lavoro relative al termine di 60 giorni per l'impugnazione del licenziamento sia prorogata al 31 dicembre 2011. È certamente apprezzabile l'accoglimento di questo emendamento perché riapre i termini per il ricorso dei precari. Ciò comporta che per tutto quest'anno non si applicherà la norma del collegato lavoro che fissava al 23 gennaio i nuovi termini per l'impugnazione dei licenziamenti. Finalmente, si riuscirà così ad approvare, per la prima volta in questa legislatura, una norma che tutela chi lavora anziché tagliare le tutele vigenti. di un fatto apprezzabile, ma non sufficiente a colmare le lacune presenti anche in questo provvedimento sul versante sociale, in particolare su quello Mi riferisco, anzitutto, al fatto che le misure a sostegno delle famiglie si presentano come disorganiche, misure tampone, molto ambiziose nell'enunciazione ma non in grado di aiutare le famiglie stesse, oggi alle prese con una crisi economica che ha determinato una riduzione del reddito a loro disposizione. Mi riferisco, inoltre, alla materia degli ammortizzatori sociali. La proroga concerne la possibilità, prevista per il biennio 2009-2010, che le risorse in materia di ammortizzatori sociali in deroga siano impiegate anche per incrementare le misure di alcune fattispecie di indennità di disoccupazione, nonché degli ammortizzatori sperimentali relativi agli apprendisti. Inoltre, la stessa proroga riguarda la possibilità di emanare decreti ministeriali per introdurre disposizioni transitorie di deroga a singole norme concernenti gli ammortizzatori sociali di specifici settori. Ho voluto citare le due deroghe perché si tratta sicuramente di possibilità di deroga positiva, ma che in questo caso si traducono in misure assolutamente insufficienti a fronteggiare la grave emergenza occupazionale presente oggi nel Paese. Un'emergenza così grave che da tempo e da più parti (ricordo in particolare le ripetute sollecitazioni da parte del governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi) si chiede la messa in campo di una riforma organica degli ammortizzatori capace di tutelare l'insieme del mondo del lavoro. Una tutela che oggi non comprende circa 1.600.000 lavoratori,

mi chiedo perché non è stato accolto un nostro emendamento che propone la modifica dei termini per la cassa integrazione straordinaria, che oggi sta sostituendo quella ordinaria. In realtà questo Governo anche su questo versante vive alla giornata e spera che la ripresa dell'economia sia tale da riassorbire i lavoratori oggi posti in cassa integrazione. Ma questo sarà difficilmente possibile perché, come sostengono quasi tutti gli economisti, siamo in presenza di una ripresa economica, peraltro molto

senza nessunissima occupazione. Ecco perché ci vuole subito una riforma organica degli ammortizzatori sociali; soprattutto una riforma che sia in grado di garantire almeno il sostegno dei redditi. Un'altra importante questione sociale che pure viene ignorata attiene alle ricadute delle modifiche introdotte dalla legge n. 122 di conversione del decreto-legge n. 78 del 2010 a carico dei lavoratori dei comparti telefonico ed elettrico. Modifiche che hanno comportato oneri rilevanti per i lavoratori iscritti ai fondi di previdenza elettrico e telefonico. Modifiche che intervengono, inoltre, negativamente

hanno avuto queste sigle sindacali in questi ultimi cinque mesi è stata sostanzialmente di latitanza. Il Governo infatti non ha saputo organizzare un incontro ufficiale con le parti sociali per affrontare il problema e scongiurare un ampio contenzioso legale in materia. Manca infine, signora Presidente, qualsiasi attenzione nei confronti dei lavoratori precari della pubblica amministrazione, settore nel quale la scadenza dei contratti a termine rischia di provocare licenziamenti in massa. Anche in questo caso, si parla di migliaia di lavoratori: chi conosce esattamente il settore parla di circa 100.000 lavoratori. Per tutte le ragioni

questa specificità, così strana eppure così condivisa. Quando si parla di montagna si immagina - almeno lo immaginano coloro che non vivono in montagna - una minoranza sperduta fra i cocuzzoli delle montagne intenti

cento del territorio complessivo del nostro Paese può essere considerato territorio di montagna in cui vive il 18 per cento dei cittadini, quindi circa 12 milioni di persone e si tratta - in questa sede può essere

attivano questa *lobby* ogni volta che c'è l'opportunità di farlo ma, come dicevo in apertura, troppo raramente. E in questi casi, purtroppo, la rivendicazione assume fatalmente l'accento del pianto, un pianto che dura da molto tempo a causa delle risposte che di Governo in Governo, di colore in colore, non si riescono ad avere. Questo, anche se negli ultimi tempi si era raggiunta una specie di intesa perfino nella definizione di montagna, una diatriba in piedi da moltissimi anni e nella quale ultimamente si sono aggiunti ai soliti parametri legati all'altitudine anche altri altri parametri condivisi legati alla situazione socioeconomica e geopolitica. Oggi saremmo in grado di definire quali sono le zone di montagna alle quali destinare le risorse specifiche. Peccato che queste risorse, di anno in anno, di legislatura in legislatura, diventino sempre più fatiscenti. Oggi si parla di federalismo: ebbene, io credo che non potrà mai nascere un federalismo autentico se non porta con sé anche un federalismo della montagna; consegnare, a chi abita in montagna, gli strumenti per gestire il proprio destino. E che questi abitanti siano capaci di gestire risorse e destino lo hanno dimostrato anche recentemente quando, sempre sotto la spinta del gruppo di parlamentari «Amici della montagna», sia alla Camera sia al Senato e questa volta in particolare al Senato, hanno dato un esempio di sagacia e capacità nella gestione delle risorse derivanti dall'industria idroelettrica. L'anno scorso, infatti, sono state redistribuite le risorse prelevate da questo settore come sovracanone idroelettrico destinato ai Comuni e ai bacini imbriferi montani, rimasto fermo per molto, molto molto tempo e rivalutato, lo debbo riconoscere e lo faccio volentieri, grazie all'impegno particolare del collega Zanetta, uno dei vice presidenti del gruppo di parlamentari «Amici della montagna».

Quando dalla montagna venivano richiesti interventi particolari, specifici, dettati proprio da questa parola, dalla specificità della montagna, molti si opponevano, il legislatore lo doveva fare: non si può, l'Europa apre una procedura di infrazione perché ogni finanziamento in più rappresenta un aiuto di Stato. Ebbene, nel Trattato di Lisbona le zone di montagna oggi sono

che ha un connotato sportivamente magari non molto rilevante ma che rappresenta ormai da un paio d'anni l'occasione per un confronto con questi due Ministri. concordato sulla necessità di spingere di più verso il riconoscimento della specificità della montagna, attraverso il riconoscimento delle peculiarità della vita, a partire dalle cose più semplici. Sono nate recentemente, per esempio, alcuni tentativi di università della montagna: penso a quella di Edro, ma anche a quella di San Michele all'Adige. Poi ci sono gli antichi negozi di vicinato, che soddisfano esigenze non solo mercantili, ma soprattutto sociali. Ci sono i prodotti tipici: altro che prodotti di nicchia! Oggi i prodotti di montagna hanno un'alta qualificazione sul mercato e andrebbero solo valorizzati e meglio distribuiti. C'è l'utilizzo delle biomasse e di tutte le altre fonti di energia alternativa che in montagna potrebbero essere addirittura esaltate rispetto ad altre zone. Vi sono poi le professioni di montagna da valorizzare:

Ma depresse da che cosa? Svantaggiate rispetto a chi? La montagna è invece un sistema perfetto, completo di risorse, di energie sotto il profilo economico, naturalistico, culturale, storico, imprenditoriale. La montagna poi ha una ricchezza su tutte: i montanari. Affinché questi ultimi possano continuare a vivere nella loro montagna dove sono nati, c'è bisogno - lì sì - di un aiuto in più, di un incentivo per dare loro ragione per rimanere lassù una vita dignitosa pari almeno a quella che avrebbero andando a cercare un'alternativa in pianura o nelle città. Non si chiede di più, non si chiedono privilegi. Si tratta veramente di un tema di pari opportunità: si vuole continuare a vivere dove si è nati, ma con una vita dignitosa pari a quella di chi poi viene durante l'estate o l'inverno come turista, ossia i cittadini, i quali non capiscono che se loro godono di ricchezze che noi gentilmente mettiamo loro a disposizione, è perché queste ricchezze sono mantenute e conservate con il frutto del nostro lavoro. C'è anche bisogno di un'altra iniziativa: unire la montagna alle città. È perfino banale ricordare in questa sede come la sicurezza della pianura nasca in montagna, come si possano evitare soltanto con opere idrogeologiche importanti in montagna i pericoli di alluvioni in pianura. C'è anche un pericolo che oggi

da respingere con tutta la forza possibile. C'è un'omologazione di ruoli, soprattutto di valori, che non possiamo accettare. Sui tagli fatti all'economia della montagna, sulla gestione dei piccoli Comuni, sugli aspetti fiscali, parlerà domani il collega Zanetta, che è molto, molto più bravo di me in queste cose, però esistono seri problemi e lo dirà in maniera esplicita. Chiudo soltanto con una citazione che riguarda il nostro romantico tentativo di inserire alcune misure per la montagna. Guardo con l'occhio umido i due relatori, che colpa non hanno. Potrei prendermela con il Presidente della Commissione bilancio. Avevamo presentato otto emendamenti, signora Presidente. Se potessi usare un'allegoria, una metafora di tipo montanaro, rapportando questa iniziativa ad una spedizione, direi: otto partiti, nessun superstite. Al massimo, un invalido, vale a dire l'ultimo emendamento, trasformato in un ordine del giorno. Erano temi di vitale importanza: la defiscalizzazione; gli aiuti per chi non ha il metano, quindi deve acquistare il gasolio; il CAI, che va difeso come azienda, come ente non economico, capace di mantenersi. È un pianto su tutti, mi sento di fare. Un anno fa qui, signor Sottosegretario, durante la discussione della legge comunitaria, in un momento particolarmente doloroso, con molte vittime in montagna sotto le valanghe, eravamo riusciti ad avere dal Governo 250.000 euro per pagare le polizze di assicurazione dei volontari - sottolineo: volontari - del Corpo del Soccorso alpino, i quali andavano fino ad allora a rischiare la vita - e molti ce l'hanno rimessa - senza nemmeno una polizza di copertura. Purtroppo, con amarezza, pur essendo il mio Governo amico, devo constatare che da domani questo succederà ancora.

Democratico, questa possibilità ora viene offerta fino al 31 dicembre del 2012. In questo senso abbiamo forse dato la possibilità ai Comuni di programmare i bilanci per quest'anno e anche per il prossimo. Qual è la cosa grave? nel decreto milleproroghe una proposta che, dal mio punto di vista, non è un segnale di buona amministrazione e di buona gestione del denaro pubblico, nel senso che quando i comuni sono costretti ad utilizzare gli oneri di urbanizzazione per fare il bilancio, per fare spesa corrente, qualcosa non funziona. Gli oneri di urbanizzazione dovrebbero essere utilizzati per fare opere di urbanizzazione primaria e opere di urbanizzazione secondaria, strade, scuole, uffici pubblici, fabbricati di questo tipo. Al limite, le manutenzioni. In realtà cosa abbiamo fatto in questi anni? Cosa avete fatto in questi anni? Avete strozzato i Comuni.

il pagamento del personale. Questo è uno degli elementi fondamentali della finanza locale. Ma in questi anni si è tagliato e dall'altra parte si è data la possibilità di ricorrere a questa «riduzione del danno» rispetto alla mancata disponibilità di risorse. Qual è la situazione oggi che hanno i nostri Comuni? Mi dispiace che in un momento in cui da una parte si racconta che si vuole dare più autonomia e che col federalismo risolveremo tutto, nella realtà stiamo togliendo loro risorse ed autonomia. Qualcuno dice con gli *slogan*: padroni a casa nostra. In realtà oggi i Comuni sono commissariati dal Ministero dell'economia. Col Patto di stabilità abbiamo tentato di fare degli emendamenti per tentare di

Ma non chiede ai Comuni il rispetto di queste norme. È il Governo italiano, il Ministero dell'economia italiano che chiede ai Comuni quello che non riesce a far fare alle altre parti della pubblica amministrazione, perché i Comuni non possono produrre *deficit*.

loro gli oneri di urbanizzazione per pagare il personale invece di fare le opere infrastrutturali e, di conseguenza, per fare le opere infrastrutturali andiamo ad aumentare l'indebitamento. Altra cosa importante: famiglie e imprese. Obblighiamo gli enti locali a non pagare i fornitori. Ossia, per rispettare il Patto di stabilità hanno i soldi in cassa, iniziano da luglio nei vari uffici comunali a chiamare le imprese e a dire: vi pagheremo a gennaio dell'anno prossimo perché dobbiamo scavallare il 31 dicembre per riuscire a dimostrare che rispettiamo il Patto di stabilità. Questo è il modo per aiutare le imprese? gli enti che hanno delle risorse proprie, che hanno saputo governare bene ed amministrare bene le proprie risorse, alla fine quei soldi devono essere "accantonati", devono produrre avanzi di amministrazione per compensare altre amministrazioni dello Stato e non amministrazioni locali, perché queste ultime non possono fare *deficit* ma possono solo fare avanzo se rispettano le norme. Ebbene, questo meccanismo perverso ha creato questa situazione:

Quando affrontiamo le norme europee diciamo che bisogna pagare a 60 giorni, e poi facciamo il Patto di stabilità che di fatto obbliga gli enti locali e territoriali a pagare nell'anno successivo per scavallare la fine dell'anno. Ecco, credo che questa sia la situazione su cui su cui probabilmente questo decreto meritava di essere valutato in modo completamente diverso. Lo stesso per quanto riguarda le famiglie, perché, ovviamente, nel momento in cui

anche quest'anno si consuma il rito del milleproroghe; un rito tutto nostro, italiano possiamo dire. Il decreto-legge, come al solito, si caratterizza per la presenza di luci e ombre. Il problema è, secondo me, che anche le luci presentano grandissime ombre per quello che riguarda il finanziamento. Le misure che esso contiene - anche questo è un dato ormai impresso nella tradizione - sono molto eterogenee tra loro, e ciascuna meriterebbe un attento esame e una valutazione caso per caso. Mi limiterò solo ad alcune osservazioni sui contenuti secondo me più importanti e di rilievo del decreto. Le proroghe non onerose, contemplate in un elenco richiamato al comma 1 dell'articolo 1, sono circa 70 e differiscono i relativi termini al 31 marzo 2011, cosa singolare, visto che generalmente il differimento è sempre stato di un anno.

Tale norma, come è stato fatto rilevare anche da alcuni colleghi senatori nelle questioni pregiudiziali, presenta dei profili giuridici abbastanza singolari. Anche a nostro avviso, essa risulta, infatti, quanto meno *sui generis*. generis*. Negli anni passati era il Parlamento, in sede di conversione, ad avere l'ultima parola sulla concessione del differimento dei termini. Nel provvedimento in esame quest'anno il Governo, dopo aver differito per un solo trimestre i termini in scadenza a fine 2010, decide di mantenere per sé la facoltà di prorogare ulteriormente gli stessi termini fino al 2011. Le Commissioni riunite 1a e 5a, ,con un emendamento, hanno mitigato quello che a prima vista è un vero e proprio arbitrio che il Governo si è autoconcesso. Le Commissioni hanno infatti stabilito, a nostro avviso in modo più logico e corretto, che ogni ulteriore proroga decisa dal Governo dovrà essere sottoposta al parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle altre Commissioni per gli eventuali risvolti di carattere finanziario. prevede anche un'altra serie di proroghe importanti sotto il profilo sia sociale che economico che comportano oneri per lo Stato. Interveniamo in tutti quei territori che hanno avuto problemi di calamità naturali differendo dal 21 dicembre 2010 al 30 giugno 2011 i versamenti per gli abitanti dei vari territori colpiti dalle alluvioni dell'inizio dell'inverno. Si tratta di un intervento di proroga importante perché riguarda il versamento di tasse, imposte, contributi previdenziali e assistenziali e premi obbligatori per le assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali; un provvedimento che comporta un impegno finanziario complessivo di oltre 90 milioni. Vi è poi tutta una serie di altri interventi con la copertura, e qui secondo me cominciamo a riscontrare numerose situazioni che vanno al di là del semplice intervento del milleproroghe, ma riguardano complessivamente la politica economica che si è attuata in questi anni. Iniziamo con l'intervento sul 5 per mille, le cui risorse ammontano a complessivi 400 milioni di euro. Il Governo mantiene la promessa che ci era stata fatta qualche mese orsono di

Vorrei ricordare che il Gruppo di Futuro e Libertà, in sede di approvazione della legge di stabilità, sia con propri emendamenti sia con ordini del giorno, aveva contribuito a far assumere al Governo l'impegno al reintegro delle risorse con un successivo provvedimento,

del Governo in sede di copertura, altri interventi che vengono messi nel milleproroghe con i soliti tagli orizzontali che, colpendo nel mucchio, colpiscono anche voci di spesa che sono indispensabili per il mantenimento e il buon funzionamento dello Stato. Stato. Una parte cospicua della copertura è caduta sulle risorse disponibili relative ai rimborsi e alle compensazioni d'imposta, che già rappresentano un problema perché ci sono grandissimi ritardi per quanto riguarda le compensazioni e i rimborsi a chi effettivamente ha il diritto di riceverli. Questi mancati rimborsi di imposta, in un momento di grande crisi di liquidità delle aziende, colpiscono proprio il mondo delle piccole e medie imprese. Il resto della copertura cade poi su capitoli quali il fondo per la finanza di impresa, i contributi all'editoria - copertura poi che è stata cambiata durante l'esame delle Commissioni - e il fondo creato dal decreto-legge n. 78 del 2010 per agevolare i piani di rientro dei Comuni commissariati, al quale vengono tolti 50 milioni nel 2011 e 24 milioni nel 2012. Vorrei ricordare altri provvedimenti, se mi è consentito, iniziando dai dai 500 milioni che vengono concessi per Roma Capitale. È un provvedimento di un certo peso, perché pone a carico del bilancio dello Stato l'onere per l'estinzione delle anticipazioni di tesoreria della Pur non volendo negare che il riequilibrio dei conti della Capitale d'Italia è una questione di primaria importanza e, al di là del fatto che il provvedimento non comporta oneri in termini di indebitamento netto ma soltanto di saldo netto da finanziare, non si può negare - dobbiamo dirlo con forza - che l'impostazione di operazioni così importanti richiederebbe una maggiore trasparenza nei confronti dei cittadini e di tutti i contribuenti italiani. Non deve infatti sfuggire a nessuno

agli impegni che abbiamo nei confronti dei tanti cittadini e delle tante famiglie che non riescono a dare un futuro ai propri figli, e pensiamo a quello che è successo, alle modalità di assunzione, ai ruoli che tanta ai ruoli che tanta gente va a ricoprire all'interno delle municipalizzate, che prendono i soldi di tutti i contribuenti, in maniera irregolare, immotivata, non giusta e non corretta.

Guardate, lo dico sinceramente e me ne assumo la responsabilità: non ero molto d'accordo quando la mia parte politica chiese le dimissioni del ministro Bondi. Ero alquanto perplesso, perché comunque, in un momento abbastanza difficile per l'economia italiana, si poteva ragionare su tutto; la cultura però rappresenta una delle nostre principali fonti di introito per quanto riguarda le casse dello Stato con il turismo. Per cui tagliare quella parte di finanziamenti che riguardavano il nostro tesoro, il nostro petrolio, il nostro patrimonio culturale non è stata una scelta di grande perspicacia e di grande progettualità. Il ministro Bondi probabilmente è stato debole nei confronti del Ministero dell'economia, ma, dopo quello che è successo, aveva preso degli impegni precisi nei confronti dei lavoratori dello spettacolo.

abbiamo lasciato il reintegro del fondo, circa 150 milioni di euro, a una tassa di scopo: un euro a biglietto che verrà pagato dai cittadini.

Poteva venire qui a difendere quello che aveva promesso ai lavoratori dello spettacolo, insieme a noi che abbiamo cercato in qualche modo di incrementare i fondi destinati a quel settore. Un'altra iniziativa profondamente iniqua,

l'ennesimo *spot* elettorale privo di qualsiasi tema di sviluppo economico, sociale, culturale od occupazionale. L'ennesimo *spot* elettorale che serve

Gli altri enti lirici, le altre fondazioni possono anche chiudere, non c'è alcun tipo di problema perché questa è la precisa indicazione del Governo emersa nel corso dell'esame del milleproroghe.

Lo scandalo vero, serio, quello che ci deve far pensare e riflettere a fondo, al di là dei

emendamenti con i quali si riconoscevano incentivi agli allevatori seri, ad allevatori che lavorano, che pagano le tasse, che se sbagliano pagano anche le multe.

Ci sarà il nuovo Patto, la legge di stabilità europea, saranno momenti molto duri. Speriamo che si possa avviare una riforma vera, che si smetta di coprire i buchi con toppe,

le confesso che mi sarebbe piaciuto poter discettare su questo provvedimento con una disponibilità di tempo almeno congrua per evidenziare alcuni aspetti che considero particolarmente gravi. Mio malgrado, dovrò limitarmi a considerazioni che rischiano di sembrare più delle affermazioni didascaliche, quasi degli slogan, piuttosto che considerazioni supportate da valutazioni puntuali e precise. Ho cercato di dare un abito a questo provvedimento e mi è venuto in mente di definirlo relativamente ad alcuni aspetti che lo caratterizzano. Signora Presidente, in questo provvedimento ci sono norme intruse, ovverosia riferimenti legislativi, proposte di tipo legislativo che non potrebbero esserci. Ci sono gravi omissioni, cioè mancano disposizioni che, viceversa, avrebbero dovuto esserci. Ci sono procedure illegittime:

Complessivamente, potremmo dire che stiamo assistendo a ciclopiche contraddizioni, a nuovi giochi di prestigio. È su un aspetto, però, che vorrei richiamare la vostra attenzione: sugli accanimenti sofisticati che si stanno consumando anche in questa circostanza. Qual è il settore, signora Presidente, colleghi, che per l'ennesima volta viene posto sotto tiro da questo Governo? Governo? Potrei dire che uno dei settori particolarmente martoriato e ferito da questo Governo è quello della pubblica amministrazione. Le gigantesche riforme del ministro Brunetta di fatto hanno dimostrato di non essere tali in quanto a dimensioni e di avere nella loro forma ridotta, viceversa, i piedi d'argilla. Fondamentalmente, il ministro Brunetta ha soltanto cercato di ottenere la benevolenza degli italiani criminalizzando la pubblica amministrazione; ha cercato di costruirsi un'immagine definendo in maniera sconsiderata, generica, *erga omnes*, un settore così delicato, che - lo ricordo per l'ennesima volta - la Costituzione considera essere apparato servente dello Stato, come un coacervo di nullafacenti, come un'accolita di incapaci, come una genia di mangiapane a tradimento. E magari, nello stesso tempo, ha cercato di far passare l'idea secondo cui questo Governo, lo stesso del quale lui - ahinoi - è elemento di rappresentanza, si occupa della sicurezza e della difesa. Signora Presidente, è scandaloso che questo Governo abbia vinto le elezioni tre anni fa lucrando sui timori degli italiani relativamente alla sicurezza ed è altrettanto scandaloso che questo sentimento, che non è soltanto la proiezione e la manifestazione di un bisogno di ordinaria tranquillità, sia stato innervato e attraversato anche da sentimenti di patriottismo. «I nostri ragazzi», dice pomposamente il ministro La Russa quando non trova manifestazioni diverse per nascondere la propria propensione a digrignare i denti. E per i nostri ragazzi, e per le donne e per gli uomini che sono preposti ad occuparsi di sicurezza e difesa, che cosa c'è? Niente, signora Presidente. Le graduatorie sono state bloccate, così come sono state bloccate per gli insegnanti le possibilità di essere assorbiti, come si dice in gergo; magari anche per i Vigili del fuoco non sono state riconosciute. I precari debbono rimanere vita natural durante precari e magari, una volta maturata una certa anzianità di precari, debbono lasciare, pur avendo onorato il nostro Paese con più missioni all'estero, là dove di sicuro non si fanno le guerre con i proiettili di gomma. È in atto, signora Presidente (e questo decreto è uno strumento ulteriore particolarmente pericoloso), lo smantellamento della pubblica amministrazione, che passa attraverso le cose che ho cercato di indicare, che passa attraverso la mortificazione dei COCER, i comitati di rappresentanza dei militari, per i quali si chiede un'ulteriore proroga, un'ulteriore dilazione, un ulteriore allungamento per interferire ed infierire in quella che è la fisiologia ordinaria e democratica di questo pezzo così importante di Stato. La stessa cosa si fa - l'ha detto da ultimo il rappresentante del Gruppo FLI - nell'utilizzo sconsiderato dei fondi che vengono dati alla nobilissima e straordinaria città di Roma: 500 milioni, pari a cinque sesti, sottratti - in barba alla legge - dai fondi che, viceversa, in quanto provenienti dalla valorizzazione di immobili del Ministero della difesa, avrebbero dovuto essere utilizzati diversamente. Signor Presidente, colleghi, ieri un milione di donne ha gridato: «Se non ora quando?». Ritengo che dobbiamo adottare tutti questa espressione, non soltanto per la funzione liberatoria che ci asseconda e che ci suggerisce, ma anche perché, con la con la nostra ulteriore pazienza e comprensione, non intendiamo correre il rischio di sembrare complici, correre il rischio di sembrare responsabili, correre il rischio di mancare al nostro appuntamento. Signor Presidente, benvenuto. Chi l'ha preceduta è stata oltremodo paziente nel condurre i lavori, e quindi mi permetto di chiederle, come hanno fatto con successo gli altri colleghi, una deroga di trenta secondi. Lo faccio, in quanto ritengo che debba essere evidenziata, conclusivamente, la vergognosa procedura che, anche in questo caso, il Governo ritiene di portare avanti. Nessuno più di lei sa, signor Presidente, quanto sia stato mortificato il Parlamento, e per esso questo ramo, in ragione dell'abitudine a portare in questa sede i decreti-legge per un'eventuale conversione, magari per il tramite della fiducia. Nessuno meglio di lei sa, signor Presidente, quanto sia doloroso per certi versi per chi, eletto o nominato, è venuto qua con la speranza di poter fare leggi e questo non gli è dato di fare, ma il tutto diventa davvero insopportabile quando per l'ennesima volta, anziché permettere una fisiologia democratica, ci viene tappata la bocca con il sistema della fiducia.

eletta (o nominata, non lo so, il significato mi è chiaro e vi è chiaro) a questo prestigioso incarico, i miei auguri personali. Il fatto che la mia parte politica abbia ritenuto di doversi caratterizzare in un certo modo non toglie niente all'apprezzamento, alla gioia, alla soddisfazione nei confronti della sua persona, che - ne sono convinto - saprà svolgere questa funzione così alta nel migliore dei modi possibili. Buon lavoro. *(Applausi dal

100 modifiche per quattro articoli costituiscono forse - certamente vi si avvicinano - un *record* nello stravolgimento del testo di partenza. C'è stata all'inizio una scrematura nell'ammissibilità, ma le riformulazioni hanno prodotto una mostruosità che manda fuori controllo le norme già debolissime sul controllo e la riduzione della spesa pubblica. Abbiamo visto scampoli e lacerti di finanziamenti a pioggia e piogge di nuovi balzelli. Ricordo le addizionali sull'energia elettrica, sui rifiuti, sui carburanti,

della Chiesa, anche dediti ad attività commerciali. C'è un aumento netto dei costi della politica: è aumentato il numero degli assessori e dei consiglieri comunali nelle grandi città; c'è un incremento delle indennità; non ci sono i presupposti di rispetto all'articolo 77 della Costituzione. È ribaltato il rapporto tra legislazione e giurisdizione, ci sono alcuni casi estremamente gravi ed estremamente indicativi, come gli abusi in Campania. Non è una bazzecola, in questo caso vengono sospesi in una sola parte del Paese effetti di sentenze penali di condanna, anche definitive, la Consulta sarà costretta a tornare su quest'argomento. Noi continuiamo a produrre dispositivi che costringono la Consulta a riprendere posizione su questioni già individuate, fissate e sceverate. È stata approvata una norma in materia di graduatorie scolastiche che non è in linea con la sentenza n. 41 del 2011, e ancora una volta,

È stato evitato lo scorrimento di graduatorie 2001-2002 nella pubblica amministrazione per continuare invece una prassi di nomine dirigenziali senza concorso. Evidentemente, la fisiologia dello *spoils system* è penetrata proprio all'interno dei precordi del modo di fare leggi. C'è un intervento sul rapporto fra TV e giornali (che in Italia è già scandaloso, perché tutti sappiamo che, benché la legge non lo permetta, il Presidente del Consiglio ha più di un giornale di famiglia) un giornale di famiglia) che sicuramente favorirà la voracità proprietaria del Presidente del Consiglio sull'argomento, a dispregio del del conflitto d'interessi, del rispetto della concorrenza, della trasparenza degli assetti societari. Tutte materie, queste - attenzione - che sono di evidente rilevanza costituzionale e comunitaria. milleproroghe mena colpi a destra e a manca, incurante di queste incompatibilità. Ognuna delle norme che ho richiamato - ce ne sono però molte altre che i colleghi hanno elencato e, forse, nessuno di noi riuscirà a farne l'elenco completo - avrebbe meritato una questione di costituzionalità propria se fosse stata inserita fin dall'inizio nel decreto. Tali norme sono però entrate prepotentemente in seguito e le Commissioni in invece di depurare il decreto da incongruità evidenti, lo hanno vieppiù inquinato con emendamenti in materie disparate ed estranee che le Commissioni competenti non hanno neanche potuto esaminare. un vizio di origine che non può essere trascurato: il decreto-legge scade il 27 febbraio, ma si è aspettato l'11 febbraio per concludere il voto sugli emendamenti. Le Aule del Senato e della Camera dei deputati lo ricevono blindato. blindato. Facciamo poche leggi, ma le facciamo male. Le modifiche non sono subemendabili. Eccetto qualche caso, nessuno ha accolto la graziosa possibilità di subemendare quello che rimaneva.

Per risolvere i problemi di quelli che molti colleghi hanno chiamato i truffatori delle quote latte, si è deciso di far mancare i fondi alla cultura: il Fondo unico per lo spettacolo aveva ricevuto promesse fino a 150 milioni e ha avuto 15 milioni. I problemi dei precari della sanità, della scuola e della pubblica amministrazione sono stati completamente dimenticati e affossati. Sono stati negati gli spiccioli necessari ai Vigili del fuoco. Parlavo ieri, in piazza, con un vigile del fuoco che mi spiegava che nella mia città, in una postazione specifica di pronto intervento, dieci anni fa erano in 21 e ora sono in Non viene pagato loro alcun straordinario; i precari sono tenuti a bacchetta, non possono protestare e sono costretti a lavorare per un salario insufficiente. Sono stati negati i soldi necessari ad affrontare il rischio idrogeologico. A tale proposito, si aprirebbe un capitolo penoso perché l'Italia è un territorio complicato, sofisticato e difficile, che avrebbe bisogno di fondi cospicui e decisivi

Nell'elenco degli argomenti che avrebbero dovuto essere riconsegnati alle Commissioni competenti si trova, per esempio, la trasmissione di informazioni su trattamenti di procreazione assistita. Viene da pensare che chi straparla di *privacy*, poi fa il contrario quando deve esercitare - chissà - forse una censura occhiuta e preventiva su cose che si ritiene dispiacciano Oltretevere. scorporo di BancoPosta da Poste italiane e la possibilità di acquisto di banche da parte di Poste: non sono esperto della materia, ma l'altro giorno, nelle Commissioni 1a e 5a riunite, ho assistito allibito ad uno scampolo di discussione quasi amichevole su questo argomento, come se si potesse decidere di cose di queste entità e peso ragionando semplicemente su un emendamento presentato all'ultimo momento. modifiche clientelari e microterritoriali oscurano le pochissime cose buone che stanno dentro il provvedimento. Il testo firmato dal Presidente della Repubblica è stato del tutto stravolto ed è diventato una sorta di finanziaria *omnibus,* che contiene spese preelettorali, non rispetta l'articolo 81 della Costituzione, viola i vincoli di contabilità pubblica che le leggi nn. 468 del 1978 e

In questo caso, penso che la Presidenza del Senato dovrebbe operare un severo vaglio di ammissibilità, escludendo tutte quelle parti che non sono in linea con il titolo, non rispondono ai requisiti di necessità e urgenza previsti dalla Costituzione,

del resto, non è una novità. Infatti, in tutti i provvedimenti di carattere generale con ripercussioni finanziarie di questa legislatura, il settore primario è costantemente risultato residuale, le sporadiche misure inefficaci e l'individuazione delle priorità incoerenti ed incongruenti. Si può dire che anche i contenuti, la forma e la procedura di questo decreto-legge rappresentino l'icona finale dell'involuzione progressiva delle politiche agricole a cui si è assistito nel corso di questa legislatura. Se si avesse voglia di ironizzare - anche se non se ne ha - si

perché da prorogare c'è rimasto ben poco: in 30 mesi sono state di fatto azzerate buona parte delle misure che avevano sostenuto il settore negli anni precedenti. Se poi si guardasse il carattere di urgenza, il sarcasmo troverebbe un terreno fertilissimo. Da mesi, infatti, vengono denunciati stati di emergenza in interi settori, che poi nelle dichiarazioni hanno sempre trovato una comprensione verbale tra i membri del Governo. Ne cito alcune. In merito alle aziende che producono in serra, l'esplosione dei costi di produzione e, tra questi, del gasolio per il riscaldamento, ha messo in ginocchio il settore. Da mesi viene richiesto il rinnovo dell'accisa a livello minimo, visto che l'esenzione prevista in altri Paesi dell'Europa ai produttori italiani non è riconosciuta, perché la procedura non si è mai conclusa e le aziende sono a rischio chiusura. al settore bieticolo, per esso si è assistito ad un'altalena di dichiarazioni, smentite e misure per recuperare, di fatto, gli 86 milioni di euro, che rappresentano la quota nazionale dell'OCM zuccheri sottoscritta nel 2005 da questa maggioranza. Nominalmente le risorse sembravano recuperate. Fu uno degli ultimi atti propagandistici del ministro Zaia, che dichiarò di aver lottato con tutte le forze per rendere disponibili almeno 21 degli 86 milioni di euro mancanti al settore. Se oggi non si interviene, le risorse già teoricamente disponibili presso l'AGEA, non potranno essere utilizzate. Inoltre, in questo provvedimento si azzera il fondo per le APA. A fronte di tanta demagogia sull'importanza di garantire la salubrità delle produzioni, questo fondo rappresentava uno dei pochi esempi di successo, che ha anche incentivato la diffusione della qualità delle nostre produzione zootecniche. Dal 1°gennaio non è più finanziato e non si è neppure cercato di immaginare un programma di razionalizzazione. Nella legge di stabilità se ne è decretata l'estinzione.

una riduzione del fatturato pari al 25 per cento, un crollo dei livelli occupazionali pari a 17.000 posti di lavoro (passando da circa 46.000 un incremento del 240 per cento dei prezzi del carburante, incidendo sui costi di produzione fino al 60 per cento per il sistema più colpito, quello della pesca a strascico. La dotazione di parte corrente per l'economia ittica è passata da 14 milioni di euro a 6 milioni. Più in generale, si può dire che per l'agricoltura, che solo nell'ultimo anno ha visto la chiusura di ben 25.000 aziende e che continua a subire sia gli effetti dell'instabilità dei mercati e della variabilità dei prezzi che il costante e inarrestabile aumento dei costi produttivi, contributivi e burocratici, l'unica e autentica emergenza è la scadenza delle rate degli splafonatori "recidivi" delle multe delle Si tratta di una manciata di aziende rispetto alle migliaia che hanno continuato a pagare e rispetto alla quale si continua a trovare un'insopportabile, inspiegabile ed ingiusta sponda nei parlamentari della Lega. Ma è possibile che, ancora una volta, l'unico argomento che esce alla ribalta della cronaca per il settore agricolo siano le quote latte? Credo si possa dire ormai che siano il simbolo delle contraddizioni politiche di questa maggioranza. In Commissione è stato presentato l'emendamento per la proroga delle scadenze relative e, mentre il Ministro comunicava ai membri della Commissione stessa un parere fortemente contrario, il rappresentante del Governo dava l'ok. l'ok. È una situazione che abbiamo già visto in precedenza, con la sola differenza che la volta precedente il Ministro aveva minacciato le dimissioni alla fine, questo è l'unico emendamento oneroso approvato per il settore agricolo. E con quale copertura? Il senatore Morando per primo, ma tutti gli interventi successivi, hanno descritto dettagliatamente dove si dove si vanno a trarre le risorse. È chiaro da questa rappresentazione che la questione non è solo agricola. Non a caso, nella quasi totalità degli interventi dei senatori che mi hanno preceduto, stato citato questo emendamento senza mai indicarlo come intervento riguardante il settore primario. Come pure è politica la questione che il Ministro, a copertura dell'assenza assoluta di interventi, tuoni che questo non è il provvedimento adatto per affrontare le gravi difficoltà contingenti e strutturali del settore. Credo sia giusto informarlo che dovrebbe andare a verificare da quanti mesi questo Senato presenta ordini del giorno, risoluzioni, proposte, molto spesso sottoscritte in modo trasversale tra tutte le forze politiche, molte delle quali hanno ottenuto un impegno a provvedere da parte del Governo appena fosse stato possibile. Ma, evidentemente, non è mai possibile: evidentemente non è mai il tempo per l'agricoltura.

Presidente, il mio intervento sarà brevissimo. L'esigenza di parlare mi viene dettata dalle ansie e dalle preoccupazioni diffusesi tra i dipendenti della Finmek di Caserta. Faccio riferimento in particolare

al termine di scadenza il programma non risulti completato il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, può disporre la proroga del termine del programma per i gruppi industriali con imprese o unità lavorative nella Regione Abruzzo, fino al 30 giugno 2011. Il riferimento alla Regione Abruzzo era stato evidentemente male interpretato, nel senso che si riteneva e si ritiene, ma a mio avviso ciò è assolutamente infondato, che il provvedimento sia applicabile solamente ai dipendenti degli stabilimenti che hanno sede in Abruzzo. Così evidentemente non è, perché il riferimento è al gruppo industriale. Non solo: c'è un precedente autorevole, vale a dire l'articolo 39 della legge 30

di preoccupazioni ed ansie che non trovano giustificazione, probabilmente alimentate anche da notizie di stampa e da qualche comunicato degli esponenti dell'opposizione che hanno ingenerato un timore che non va assolutamente condiviso.

Vorrei precisare che si tratta di un problema complesso e difficile, che riguarda 60.000 abitazioni. Il tutto è stato ulteriormente esacerbato da una dichiarazione di incostituzionalità di una norma regionale fatta fatta improvvidamente dalla Giunta Bassolino, che non ha dato la possibilità ai proprietari di quelle unità abitative di poter condonare. Questa pausa di riflessione servirà sicuramente, dal momento che la Regione Campania ha emanato il piano casa e dovrà emanare un piano paesaggistico. Distruggere 60.000 abitazioni non è impresa da poco; non solo, c'era anche la sperequazione che si era creata tra coloro che subivano l'abbattimento rispetto

il riemergere di quelle preoccupazioni di ordine sociale e di ordine pubblico che si stavano consumando sul territorio della Campania. Signor

aumentata ed alimentata, qualora ne dovessero ricorrere le condizioni, con un provvedimento amministrativo da parte del Ministro del lavoro. Signor Presidente, il decreto milleproroghe e la sua conversione in legge di cui oggi si dibatte poteva essere un'occasione con cui la maggioranza poteva rimediare alla stasi che il Governo ha imposto ormai da troppo tempo, coinvolgendo i suoi rappresentanti nelle Aule parlamentari. In un contesto sociale in cui la crisi è dominante, l'attività parlamentare avrebbe dovuto essere proficua e dominante. Ciò che i cittadini chiedono alla politica è che sia vicina ai loro problemi e che li affronti nel migliore dei modi. Se poi ci riferiamo a chi è stato scelto per rappresentarli, per questi diventa un dovere. Ho fatto questa breve premessa, perché vorrei sollecitare una riflessione da parte di tutti. A fronte di provvedimenti che vanno discussi con una connotazione prettamente politica, e quindi ognuno è legittimato nelle proprie scelte, ve ne sono altri che non possono avere una collocazione politica, uno schieramento piuttosto che un altro: sono i provvedimenti che devono essere affrontati

ma abbiamo esteso il nostro intervento anche alle disabilità gravi, argomenti sui quali non esiste l'idea o il presunto dovere di fare scelte politiche. Non è necessario e non occorre ricercare una collocazione, di destra, di sinistra, di centro, quella che sia. In questo caso dobbiamo essere guidati solo dalla nostra coscienza, dalla nostra dignità di cittadini italiani, prima, e di parlamentari, poi. Non vi può e non vi deve essere demagogia là dove vi sono persone che soffrono e, con loro, intere famiglie. Pertanto, invito ciascuno di voi a vivere almeno un giorno insieme ad una di queste persone, ad una di queste famiglie. Allora, solo allora, si potrà capire di cosa stiamo parlando e quanto sia nobile il gesto che dovremmo fare per rendere loro la vita un po' più agevole. Lo dico anche al ministro Tremonti, che non è qui con noi, ma che con i suoi tagli sta mettendo a dura prova queste famiglie. Abbiamo presentato ordini del giorno, con i quali si vuole spazzare via ogni demagogia. Semmai si chiede un approccio veramente responsabile su un argomento che, peraltro, è stato anche oggetto di una manifestazione pubblica, quanto mai sacrosanta. Era in occasione dell'approvazione del Patto di stabilità, quando il Governo destinò una quota di 100 milioni di euro per i malati di SLA e per le loro famiglie. Chiedo a lei, senatore Malan, che ritengo una persona veramente sensibile:

non si può lesinare su questi interventi finanziari. Inoltre, è inconcepibile che non vengano prese in considerazione anche altre disabilità gravi, gravissime. Si chiede che questi finanziamenti siano destinati ad interventi per ricerca e assistenza domiciliare, sia per i malati di SLA sia per tutti i malati con gravi disabilità: una quota non aggiuntiva rispetto alle risorse stanziate per le stesse finalità della legge di stabilità 2011, trattandosi, al contrario, delle stesse risorse che concorrono alla determinazione nell'ammontare indicato. Non possiamo consentire l'azzeramento del fondo per la non autosufficienza, ossia i 400 milioni che vengono a mancare da quest'anno, e che tutto questo passi inosservato. Sostengo, e con me tutto il mio partito, ma credo anche voi, che occorra avviare un'ampia riflessione sul mondo delle patologie gravissime. Potremmo individuare misure di carattere generale,

In definitiva, è quanto mai necessario adottare un progetto condiviso, sia perché si cerca di far fronte ad un grande dramma, sia perché si incrementa la ricerca in Italia, che porterà, ne sono sicura, benefici a queste persone sfortunate e all'intera collettività. E se l'argomento dovesse ricadere sulla mancanza di risorse, allora io ribadisco che questi provvedimenti hanno una priorità assoluta

Il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. reca «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie» e adotta una tecnica legislativa nuova che differisce da quelle che hanno caratterizzato i precedenti decreti cosiddetti milleproroghe. Quei decreti, come è evidenziato anche dalla relazione tecnica del Servizio studi, hanno tradizionalmente affiancato commi che impiegavano la tecnica della novella (ossia della modifica testuale di atti legislativi previgenti) a commi che, senza modificare formalmente le disposizioni previgenti, disponevano la proroga della sua efficacia temporale. Nessuna delle due tecniche certamente è in grado di ovviare alla inevitabile mancanza di chiarezza dei testi normativi che è insita nel fatto stesso di prorogare la lettura risultava comunque agevolata grazie al fatto che i commi erano raggruppati per materie, in articoli dotati di rubrica (proroga di termini in materia di istruzione, in materia sanitaria, e via dicendo). l'articolo 1 del decreto fissa un nuovo termine per 63 disposizioni previgenti inserite in una tabella che, nella maggior parte di casi, non contiene elementi esplicativi del loro oggetto. Inoltre, l'applicazione del termine disposto dall'articolo 1 alle disposizioni elencate nella Tabella 1 implica talvolta un procedimento interpretativo dagli esiti non sempre di immediata evidenza. Non vi è dubbio che lo stesso titolo del provvedimento chiarisce che il decreto legge non si limita a prorogare termini di leggi vigenti ma inserisce nuove disposizioni in contesti normativi già vigenti o, come nel caso degli interventi di Roma Capitale, del tutto innovativi. Anche nell'amplissimo numero di leggi indicate nella tabella allegata, gli interventi previsti non si limitano alla proroga di termini, ma consentono, tramite la possibilità di intervenire sui "regimi giuridici " (come è previsto dal comma 2 dell'articolo 1), l'inserimento di innovazioni Quindi l'articolo 1, comma 2, autorizza il Governo a modificare, con una fonte secondaria, i termini di vigenza di normative contenute in fonti di rango primario, al di fuori delle procedure e delle garanzie previste per i regolamenti di

Detto questo, più che parlare di ciò che è contenuto nel decreto oggi al nostro esame, credo sia necessario evidenziare ciò che non c'è e cosa si sta cercando di far entrare nel testo proprio per quanto detto prima. Il presidente Baldassarri ha già illustrato magistralmente sia da economista che da politico i nostri emendamenti 2.1001, 2.1003 e 2.1004.

Penso ad esempio all'emendamento sulla fecondazione assistita che, di fatto, vuole schedare tutte le donne che si rivolgono ai centri italiani di procreazione medicalmente assistita e che, in un certo senso, rappresenta un ulteriore inasprimento della legge n. Con un atto di forza, utilizzando lo strumento del milleproroghe, il Governo - che non può, infatti, introdurre nuovamente i divieti che sono stati cancellati dalla Carta costituzionale nella legge n. 40 - in realtà introduce la violazione della *privacy*, creando un ulteriore deterrente all'accesso a tecniche di fecondazione. E questo è grave. L'altro punto, di cui non posso non parlare anche se è stato ampliamente oggetto degli interventi che mi hanno preceduto, è quello delle quote latte. E' stato infatti approvato in Commissione l'emendamento che rinvia di sei mesi la scadenza per coloro che hanno superato le quote consentite per Uno slittamento che comporterà oneri per circa 30 milioni per l'anno in corso: 30 milioni per pochi non in regola a fronte di molte aziende che hanno creduto nello Stato e che si sono messe in regola spesso affrontando dei sacrifici economici molto duri. Qui dobbiamo ancora una volta leggere questo modo di agire in senso politico e ancora una volta dobbiamo dire che assistiamo ad una forzatura per la sopravvivenza dell'alleanza PdL-Lega che una volta si manifesta con il voto, così come proposto dalla Lega, su un federalismo che in realtà presenta ogni volta, alzando il velo, quello che realmente è - quindi non il federalismo che tutti vogliamo e che abbiamo votato convintamente, ma spesso un finto federalismo - e una volta, invece, sul far passare un'ulteriore proroga del pagamento delle multe sulle quote latte. Il testo del milleproroghe offrirebbe un non trascurabile aggancio per intervenire sulla critica situazione degli utenti *sine titulo* degli alloggi militari. Abbiamo presentato una serie di emendamenti perché si tratta di una categoria nei confronti della quale il Ministero della difesa ha cambiato in maniera repentina e non chiara il proprio approccio proprio sul versante del diritto all'abitazione. Abbiamo presentato Abbiamo presentato un ordine del giorno con altri colleghi che è stato accolto qualche mese fa in in occasione del recente provvedimento di stabilità, ma ad oggi l'impegno del Governo non si è concretizzato. Per esempio, c'è un emendamento di particolare importanza che, riferendosi all'applicazione del canone di indennità di occupazione a carico di utenti *sine titulo*, prevede che venga prorogato il termine in cui i singoli utenti, resi edotti, con le modalità e formalità in vigore, dell'importo del nuovo canone di indennità di occupazione loro applicato manifestino una ufficiale accettazione del provvedimento. Abbiamo previsto per esempio che siano escluse dal campo di applicazione le famiglie al cui interno viva un portatore di grave handicap; abbiamo comunque agganciato tutto ciò ad una verifica di sostenibilità familiare anche sulla base del reddito della famiglia.

in occasione della manovra del luglio scorso, trasferendo all'INPDAP tutte le risorse umane, finanziarie e strutturali che facevano capo a quell'ente sulla base delle risultanze del bilancio di chiusura alla data di entrata in

dell'organo di rappresentanza, fino ad oggi eletto dagli iscritti, e quindi si voleva riconoscere con questo emendamento per gli iscritti ex ENAM di avere una propria rappresentanza elettiva all'interno dell'INPDAP. Un'altra proposta che non è stata accolta riguarda la Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, una Commissione che è, a tutti gli effetti, un'autorità amministrativa indipendente come hanno sancito alcune norme di legge che l'hanno formalmente equiparata alle altre *Authority*. La Commissione è composta di nove membri nominati dai Presidenti di Camera e Senato e si pone come fulcro del sistema per quanto concerne la disciplina in materia di sciopero, in quanto ha ampi poteri finalizzati a garantire il rispetto delle procedure previste previste dalla legge attraverso le quali si snoda tutto il procedimento pubblicistico di fronte alla Commissione, alla quale compete di stabilire se lo sciopero è legittimo o non lo è. è. Scopo della legge è quello di assicurare un giusto contemperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e il diritto dell'utenza. Il punto però è questo: la Commissione non dispone di un proprio ruolo di personale, come tutte le altre autorità amministrative indipendenti, e si avvale soltanto di un contingente di 30 unità, posto in posizione di comando o fuori ruolo da parte di altre pubbliche amministrazioni. Per questo l'emendamento era volto a garantire un efficiente ed adeguato svolgimento delle funzioni attribuite alla Commissione e a dare certezza e giusto riconoscimento al personale interno che da anni si prodiga con senso di responsabilità. Concludo ricordando due emendamenti che meraviglia non vengano accolti, soprattutto oggi, quando i dati della Banca d'Italia ci dicono che il debito pubblico è ulteriormente aumentato: un emendamento secondo me virtuoso - dichiarato oltretutto inammissibile, ma di cui voglio parlare - che si pone l'obiettivo di impedire a magistrati ordinari, amministrativi e contabili,

Per molti di questi *civil servants* - sempre gli stessi - le nomine sono vere e proprie operazioni economiche. Meraviglia e un po' insospettisce l'ostracismo dimostrato ripetutamente su questo punto, in un momento, come dicevo, di obiettiva difficoltà economica del nostro Paese. Così come stupisce che non sia stato accolto dalla Commissione bilancio un emendamento che riapre i termini per rideterminare il costo di acquisto dei terreni edifìcabili e agricoli, a beneficio di persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali che in caso di vendita avessero realizzato una plusvalenza. Meraviglia perché lo Stato incassa tasse su potenziali vendite, cioè non ancora eseguite, ovvero incassa tasse in anticipo, quindi la misura invoglia i privati a vendere i terreni e soprattutto a dichiarare il prezzo di vendita. l'erario incassa anche dal compratore un'imposta di registro, catastale ed ipotecaria pari al 11 per cento, nel caso di terreno già edificabile, e al 18 per cento, nel caso di terreno ancora agricolo ma potenzialmente edificabile.

quando la plusvalenza era soggetta ad un'imposta sostitutiva del 20 per cento e quindi molto alta. In conclusione, vorrei dire che l'auspicio più volte fatto di un confronto costruttivo - quello che noi vorremmo - tra opposizione e maggioranza, nel reale interesse del Paese, è stato nuovamente disilluso. Sappiamo, infatti, che quasi certamente sarà presentato un maxiemendamento e che sicuramente verrà chiesta per l'ennesima volta a quest'Aula la fiducia. Per l'ennesima volta, dunque, il Parlamento sarà esautorato dalla sua funzione primaria, quella legislativa. Ciò compromette pericolosamente l'equilibrio che la Costituzione disegna tra Governo e maggioranza e tra maggioranza e opposizione ed è evidente che il Governo usa impropriamente l'istituto della fiducia come strumento di controllo

con il decreto in esame ci troviamo di nuovo a dare seguito alla prassi, ormai purtroppo consolidata in questa legislatura, di esaminare una congerie di norme riunite in un contenitore *omnibus* per affrontare questioni che, al contrario, potevano essere trattate all'interno di provvedimenti organici e omogenei per materia, o ancora, nell'ambito della discussione sulla manovra di bilancio (anch'essa, comunque, da qualche tempo ridotta all'osso), senza dimenticare che lo stesso testo si presta a tentativi di integrazione che immancabilmente e naturalmente sono stati posti in essere da parte di maggioranza e opposizione. Vorrei però sottolineare come la maggioranza e il Governo ne abbiano approfittato per tentare di far passare novità normative, con dei veri e propri blitz che ci colgono di sorpresa nei contenuti, perché evidenziano un comportamento incerto o, a dir meglio, schizofrenico degli stessi che, da una parte, con pubblici proclami, dichiarano di lavorare per la crescita economica del Paese, per la libertà di impresa, l'innovazione, la ricerca e la semplificazione, dall'altra, senza dirlo ad alta voce, cercano di far passare misure che vanno esattamente nella direzione opposta. Mi riferisco, ad esempio, al tentativo sventato di tornare indietro nelle liberalizzazioni della vendita dei medicinali da banco, introdotte dal ministro Bersani del precedente Governo, ed impedire l'apertura di nuove parafarmacie, vincolando alla discrezionalità dei Comuni il trasferimento di quelle esistenti. O ancora, penso all'emendamento del Governo che fissa la tassa di un euro sul biglietto di ingresso nei cinema per finanziare gli incentivi fiscali allo stesso settore. Anche in questo caso si penalizza l'impresa determinando la contrazione dei consumi in un momento in cui occorre invece risollevare la domanda e, soprattutto, si mettono le mani nelle tasche degli italiani con una tassa a carico degli spettatori. Allo stesso modo, si mettono le mani nelle tasche degli italiani (cosa che questo Governo proclama costantemente di non voler fare) chiedendo ai cittadini e alle imprese colpiti da calamità naturali l'ulteriore sacrificio di pagare nuove tasse per la propria Regione con l'aumento delle addizionali IRAP ed IRPEF e delle accise per l'energia da parte di Comuni e Province. Si può proprio gridare che al danno e alla sofferenza si aggiungerebbe un'ulteriore punizione, questa volta inflitta dallo Stato. Sarebbero quelli descritti interventi che vanno nel senso di aiutare le imprese, il sistema produttivo, i cittadini in una contingenza caratterizzata da una crisi economica non ancora sopita? Quali norme introdurre, invece, compatibilmente con questo provvedimento per perseguire queste finalità? Magari una norma che prevede la proroga del credito di imposta in favore delle imprese per le spese sostenute per promuovere la ricerca, già introdotta dalla legge di stabilità solo per investimenti fino al 31 dicembre 2011. In realtà, si tratterebbe di una minima misura perché sappiamo che il credito di imposta introdotto con la legge finanziaria 2007 come contributo automatico commisurato ai costi sostenuti per le attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo è stato modificato in negativo da questo Governo (anche questa volta senza annunci, ma sottovoce) nell'odioso meccanismo della prenotazione obbligatoria, cosiddetto *click*, che esclude molte imprese dal beneficio sulla base di un criterio di scelta che è tutto meno che meritocratico. In un'Italia che non presenta dati incoraggianti di crescita e che investe in ricerca e sviluppo meno dell'1 per cento del PIL e in termini di innovazione e competitività è agli ultimi posti delle relative classifiche, sarebbe bene intervenire con misure significative strutturali che non abbiano una durata fugace come quella introdotta dalla legge di stabilità. Peccato che sul credito d'imposta il Governo in questo provvedimento interviene in modo ancora più pesante riducendo le somme destinate per le compensazioni che le imprese attendono invano da tempo, come anche ricordato in precedenza dal senatore Morando. Sarebbe poi stato opportuno porre rimedio alle disposizioni introdotte con la stessa legge di stabilità per l'anno in corso a carico di un settore imprenditoriale che ormai evidentemente viene considerato da sacrificare, quello delle TV locali, che con il passaggio al digitale terrestre avrebbero dovuto trovare un maggior spazio di crescita anche in conseguenza del principale obiettivo della introduzione del digitale: il pluralismo dell'informazione televisiva. Al contrario, si è penalizzata la libertà di impresa e si sono create difficoltà alle stesse imprese nel gestire la transizione in tempi ristretti e con una grave e repentina riduzione delle frequenze a disposizione. manca di coerenza nei confronti delle imprese anche nell'introdurre in questo provvedimento la norma che prevede la deduzione forfetaria per gli esercenti impianti di distribuzione dei carburanti. Infatti, si tratta di una misura utilizzata negli ultimi 15 anni che potrebbe considerarsi strutturale di per sé anche se viene annualmente rinnovata. In tal caso è stata riproposta, ma a metà, innovando *in peius* rispetto alle previsioni dei passati anni, limitandone l'applicazione senza produrre pertanto l'effetto auspicabile per i destinatari. Potremmo anche soffermarci a fare alcune considerazioni sull'approccio con cui anche in Parlamento siamo costretti ad affrontare il tema della riforma della giustizia, indispensabile per cittadini ed imprese. A causa della foga e del furore codificatorio da novello Napoleone - senza averne i presupposti - del Presidente del Consiglio, spesso si raggiungono risultati che deludono le aspettative per le difficoltà di applicazione che può portare la fretta che, come noto, è sempre cattiva consigliera. Penso, ad esempio, alla pseudoriforma del processo societario, approvato in tutta fretta dal Governo Berlusconi precedente e abrogato dall'attuale Governo perché rivelatosi un vero e proprio fallimento. E in questo provvedimento - mi riferisco alla media conciliazione - se in un primo momento si era trovata un'intesa in Commissione per ritardare l'entrata in vigore dell'istituto, forse nella consapevolezza della difficoltà legata all'immediata applicazione, all'improvviso sono cambiate le carte in tavola per far slittare di un anno l'entrata in vigore solo per il condominio e per gli incidenti stradali, perdendo l'occasione di affrontare con sistematicità il problema. In conclusione, onorevoli colleghi, vorrei ricordare a tutti noi che il Paese non si merita, né ora, né per il futuro, un Parlamento che legifera sempre e solo seguendo l'emergenza del momento, o comunque obiettivi di breve respiro e di ridotta portata. È ora che questo Governo presenti al Parlamento un programma per l'economia di medio e lungo termine per la crescita e lo sviluppo, che preveda interventi organici. Mi chiedo quanto dovremo aspettare, ad esempio, venga definito il disegno di legge sulla concorrenza che ormai da troppo tempo si rimanda, nonostante le ripetute sollecitazioni ed i richiami dell'Antitrust. Ne abbiamo bisogno per garantire mercati più aperti in favore della concorrenza e della competitività delle imprese, per superare i monopoli che ancora esistono nel nostro Paese, a tutela del cittadino consumatore che sta soffrendo degli effetti della crisi e del forte ribasso del potere d'acquisto di salari e pensioni. Il progressivo aumentare dei premi assicurativi, delle tariffe dell'energia elettrica ma, soprattutto, del gas ne sono un esempio.